Comunico che non sono pervenute designazioni per la composizione delle liste bloccate relative alle votazioni per le elezioni dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria, all'ordine del giorno della seduta odierna. Pertanto le predette votazioni avranno luogo in altra data da stabilire.

con il quale si istituisce, presso il Ministero della salute, la banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), finanziata con 5 milioni di euro. Si tratta di una banca dati nazionale nella quale ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto. si dà delega al Governo di come spendere i 5 milioni di euro stanziati. Presidente, stiamo discutendo esattamente della stessa materia. Stiamo esaminando un disegno di legge, già approvato dalla Camera, che prevede il deposito presso le strutture regionali.

salvo che il Governo non voglia presentare successivamente un decreto-legge per modificare quello che Camera e Senato hanno appena fatto. È un guazzabuglio difficilmente digeribile e credo che non serva neanche alla dignità della Camera e del Senato muoversi in questa direzione.

che ieri in Aula abbiamo respinto emendamenti relativi al registro nazionale delle DAT e che a farlo sono stati soprattutto i membri di quella maggioranza che ha approvato l'emendamento in questione ieri alla Camera. Questo mi fa pensare a un utilizzo truffaldino dei Regolamenti parlamentari. È evidente che, siccome non si vuole che il Senato modifichi in nulla questo provvedimento per evitare il rischio del suo ritorno alla Camera, si dà un colpo al cerchio e una alla botte

che travalica ampiamente il senso della nostra democrazia e piega invece a una logica di potere ben precisa quanto si è voluto fare ieri alla Camera e si vorrà fare la settimana prossima al Senato. Ne ha facoltà, senatore Quagliariello, ma mi auguro che non sia sullo stesso argomento. Non è infatti consentito dibattere sulla ammissibilità degli emendamenti al Senato. Figuriamoci se possiamo farlo rispetto all'altro ramo del Parlamento. Signor Presidente, lei ha assolutamente ragione da un punto di vista formale. Credo che ci sia lo spazio per un commento, invece, di carattere politico, perché la situazione che è stata denunciata dai colleghi che mi hanno preceduto è al limite.

è necessario forzare i Regolamenti fino a cambiarli, utilizzando provvedimenti che stanno procedendo parallelamente. Che cosa è accaduto, signor Presidente? È molto semplice. Ci si è resi conto che i registri regionali sono un controsenso fondamentalmente, si può verificare la situazione limite per la quale uno rilascia una dichiarazione in Campania e un'altra in Sicilia, Sicilia, secondo lo spirito antico del Regno delle due Sicilie dove c'erano due capitali, una a Napoli e una a Palermo. Ovviamente, questo concetto può ripetersi anche per altri Stati preunitari.

Signor Presidente, lei ha assolutamente ragione nel momento in cui dice che questo ramo del Parlamento, dal punto di vista regolamentare, non può intervenire su un emendamento che è all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Mi consenta - e consenta all'Emiciclo - di sottolineare una situazione che è un assurdo da un punto di vista legislativo. Infatti, quando i due provvedimenti verranno approvati, questi si troveranno oggettivamente in conflitto e ci sarà bisogno di un ulteriore

Comunico che sono pervenute alla Presidenza alcune richieste di votazione a scrutinio segreto. La Presidenza ritiene ammissibili le richieste riferite agli emendamenti 1.5005, 1.1742, 1.5008, 1.1748, 2.5, 2.5000, 2.65, 3.57, 3.5001, 3.5003, 3.5004, 3.120, 3.5006, 4.16, 4.5000, 4.101, 4.102, 4.5004, 4.5005, 4.386, 4.0.104 e 5.53, che attengono i diritti tutelati dagli articoli 13, 31 e 32 della Costituzione.

«I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione».

ritorna sempre il tema della vincolatività della dichiarazione, che rappresenta il nodo fondamentale e soprattutto divisivo del provvedimento Io invito tutti a riflettere circa la possibilità di un provvedimento condiviso se sciolto positivamente questo nodo, se si dovessero cioè ritenere le dichiarazioni anticipate quali orientamenti non lesivi della responsabilità finale del medico, d'intesa con i famigliari, sui trattamenti da adottare. Io penso che l'Assemblea si assuma una grave responsabilità negando questa possibilità d'intesa.

però constatare che non sono più quei tempi, se il Partito Democratico in particolare si chiude a a questa possibilità d'incontro, a questa possibilità di mediazione: viene da dire davvero che stavamo meglio quando stavamo peggio. Bei tempi quando c'era il Partito Comunista.

il medico, prima di iniziare a esercitare la sua professione, fa un giuramento e segue un codice deontologico, che all'articolo

fatto che nella vita del medico professionale non ci può essere l'accanimento terapeutico. L'articolo 4 recita che il medico, nell'esercizio della professione, deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità delle persone e, quindi, non deve solo soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la diretta responsabilità professionale ed etica del medico». Se noi vogliamo togliere qualsiasi responsabilità penale al medico e agli operatori sanitari, che non saranno perseguiti quando interrompono alimentazione e idratazione e potrebbero incorrere nel di istigazione al suicidio o aiuto al suicidio della persona, questa è la prova che si tratta comunque di un'eutanasia mascherata. Proseguo con l'articolo 16: «Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente, laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della Potrei continuare con gli articoli 33 e 35, ma cito in particolare l'articolo 38: «Il medico deve attenersi, nell'ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa».

anche perché qui sta succedendo qualcosa di veramente strano. Prima pretendiamo certificazioni su certificazioni alle professioni mediche e ai liberi professionisti e poi, a un certo punto,

una legge - e qui sembra che ce lo dimentichiamo - non ha come obiettivo logiche elettorali o di *spot*. La legge deve rispondere a precise esigenze e quando, invece di rispondervi, porta a dei problemi o addirittura a ingiustizie più profonde di quelle che dovrebbe sanare, perché la strada è spianata per questo, non fa il suo buon servizio; tantomeno

che hanno lo stesso contenuto, sono rivolti ad escludere che alla relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico contribuiscano soggetti appartenenti al personale sanitario diversi dal medico. Siamo ancora in presenza di una - non so se consapevole - volontà di delegittimazione del medico e delle caratteristiche esclusive e originali

non possa che esservi l'esclusiva competenza del medico nel dialogo ovviamente con il paziente ed i famigliari.

l'emendamento 1.1028 a mia firma, di analogo contenuto degli altri, è volto ad impedire che il medico possa svolgere qualsiasi attività di tipo eutanasico o in contrasto con la legge e con le regole Grazie che implicitamente pone l'Assemblea di fronte alla possibilità di codificare il divieto dell'eutanasia. Sarebbe davvero colpevole un voto dell'Assemblea che, invece, rigettasse questo emendamento, perché concorrerebbe ad alimentare quelle interpretazioni che conducono a ritenere il provvedimento la prima fonte regolatoria di pratiche eutanasiche, ancorché di tipo omissivo. Infatti, che «il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica». Insomma, no all'eutanasia.

con alcuni passaggi molto semplici. Il medico non può prendere in considerazione orientamenti atti a cagionare la morte del paziente.

di far sì che il paziente riesca a vivere più tempo possibile. Nel momento in cui mettiamo i medici nelle condizioni di far morire il paziente, si va contro il codice deontologico del medico.

ci sono diversi colleghi presenti in quest'Aula e sappiamo bene tutti cosa significa accanimento terapeutico e cosa - invece - significa favorire la morte di un paziente che arriva fino all'eutanasia.

e, con la grande chiarezza di dire la verità all'interno di quest'Aula, si confermi che tutto quello che hanno sostenuto i colleghi fino ad oggi corrisponde alla realtà.

Signor Presidente, nel sostenere questo emendamento, che mira a sopprimere parole relative all'eventuale rifiuto del trattamento sanitario, voglio nuovamente (lo stiamo facendo da ieri, ma il tema non è banale)

alcuni colleghi hanno richiamato l'attenzione dell'Assemblea, e anche della Presidenza e del Governo, sul modo disordinato con cui si sta procedendo, nonché sull'uso improprio del disegno di legge di bilancio in discussione alla Camera.

Abbiamo visto che questo principio è stato ripreso alla Camera, che è stata l'unica Camera in questa ultima fase legislativa perché qui stiamo respingendo in sequenza gli emendamenti; non facciamo riflessioni perché stiamo al fine vita, al fine legislatura, al fine tutto. Oggi i giornali hanno anche scritto la presunta data delle elezioni, quindi bisogna votare in maniera conforme anche laddove si dovrebbe cambiare il disegno di legge. Dopodiché, nel corso dell'esame della legge di bilancio alla Camera la Commissione affari sociali ha approvato un emendamento di Marazziti e Gelli che istituisce, presso il Ministero della salute, la banca dati,

questione alla Camera è emersa. Noi abbiamo anche rilevato come il Governo, nella persona della sottosegretaria Biondelli, abbia espresso un parere conforme alla relatrice sugli emendamenti al disegno di legge di bilancio, tranne che su quello a firma Marazziti e Gelli, rispetto al quale si è rimessa alla Commissione.

perché manca una cosa fondamentale. È corretto questo modo procedere per cui alla Camera si fa un'altra cosa? È conforme ai Regolamenti del Parlamento? Pongo quindi ulteriormente, come già altri colleghi, una questione sulla correttezza del modo di procedere nell'intreccio di questo di legge di bilancio e le norme dei Regolamenti del Senato e della Camera. Non mi pare una questione banale. Dopodiché, ho letto anch'io i giornali questa mattina che dicono che si vota il 4 marzo; a parte che non lo sappiamo perché sono altre istituzioni, che, com'è ben noto, che devono decidere, sentiti anche i Presidenti di Camera e Senato. di Camera e Senato. Essendo vice Presidente del Senato, non farò discussioni o polemiche sui ruoli politici. Anche perché io sono un politico e mi scandalizzo poco se si assumono ruoli politici. Io sono contro l'ipocrisia che vuole "asessuate" alcune figure istituzionali; siamo tutti politici, anche chi diventa Presidente di un'Assemblea. Intendo

che dovrebbe essere aggiustato in quel modo. Ma chi ce lo dice, poi, se la legge di bilancio verrà approvata effettivamente con quella norma? E poi deve tornare il Senato, perché torna al Senato. È un modo non serio, non regolare, di legiferare su questioni fondamentali. Quindi, voterò a favore di questo emendamento del collega Centinaio anche con queste ulteriori motivazioni. Le questioni che stiamo ponendo, infatti, sono queste e sono talmente fondate che anche loro alla Camera, "travestiti" da Marazziti e non potendolo fare al Senato, pongono una questione che noi abbiamo posto e alla quale ci si dice no.

questo emendamento del senatore Centinaio perché esso ripropone e riposiziona il centro di questa legge: no alla eutanasia e no all'accanimento terapeutico. Vede, signor Presidente, noi abbiamo legiferato su altri temi sensibili in quest'Aula e, anche lì dove abbiamo legiferato con maggiore puntualità,

scritta puntualmente, precisamente, e la volontà del legislatore era precisa e riconoscibile in tutte le parole della legge: eppure, la magistratura un po' alla volta l'ha smontata. Ora, io credo che qui in quest'Aula nessuno voglia l'eutanasia e l'accanimento terapeutico, ma se noi non lo scriviamo nel provvedimento, le zone d'ombra potranno rendere plausibile qualsiasi interpretazione.

sappiamo che ogni medico ha questo divieto per deontologia ma lasciamo anche questo in una zona d'ombra, perché qualcuno possa interpretarlo. possa interpretarlo. Se noi vogliamo essere dei legislatori seri, dobbiamo scrivere seriamente i nostri sì e i nostri no.

proprio perché non abbiamo voluto trattare in questo provvedimento la problematica dei registri, l'altro ramo del Parlamento sta ovviando a questa mancanza

quindi, se il percorso sui registri non verrà terminato alla Camera, noi avremo una legge monca e diritti che una parte del Parlamento vuol dare ai cittadini italiani che non saranno esigibili su tutto il territorio nazionale. *(Applausi

Secondo voi e secondo questo testo il compito del medico sarà quello di informarmi su cosa mi succederà se rifiutassi il trattamento sanitario o perfino l'accertamento diagnostico. Posso addirittura rifiutare che mi venga fatto l'accertamento diagnostico per sapere che

che queste sono le disposizioni anticipate di trattamento dell'eutanasia, almeno avreste fatto un servizio migliore al Paese; invece, ancora una volta, fate i codardi.

Come si evince dalla titolazione di questo disegno di legge, si pone, all'interno dello stesso, sia il consenso informato che le cosiddette disposizioni anticipate. Se nell'ambito del comma 3 è del tutto condivisibile che ogni persona abbia il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute, alla fine del comma 3 3 si riporta che ogni persona può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare - e qui c'è il *vulnus* - i familiari o una persona di sua fiducia incaricata di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece,

si crea una contraddizione tra l'informazione che viene data a un familiare, il consenso che viene chiesto ai familiari e il fiduciario che sarebbe singolo. Grazie delega i familiari a esprimere un consenso: un minimo di logica detta di quale conflitto si vada a creare quando siano più familiari che debbono esprimere un consenso. Ecco perché io ritengo sia corretto,

l'informazione può essere data anche ai familiari che possano tradurla - a livello linguistico, concettuale, di sensibilità e varie - al paziente, ma sarà sempre lo stesso paziente, se nel pieno delle proprie capacità, a esprimere un consenso. Mi sembra del tutto originale, sotto il profilo giuridico (e quindi, evidentemente, anche legislativo), che l'informazione la si dia ai familiari e saranno gli stessi poi a dover esprimere un consenso: no, il consenso verrà demandato a un familiare solo quando si è in condizioni di incapacità di agire, questo è il senso dell'emendamento che ho presentato. Altrimenti, si verrebbe a creare una situazione del tutto paradossale dove più familiari si sentono titolati di un rapporto fiduciario in una situazione di conflitto dove ognuno andrebbe a interpretare una verità personale mediata per un soggetto che non è capace di intendere o volere o che non sia, più

discuteranno di qual è la volontà della persona. Quindi, se ci sono il fiduciario, le dichiarazioni e quant'altro, è ovvio che ci deve essere un familiare delegato alle decisioni. Il collega Romano ha voluto prefigurare il caos che si può determinare.

non posso decrittare le loro affermazioni). Lei, senatore Romano, ha posto un problema che nel concreto si traduce nel balletto intorno al letto della persona morente con i familiari, che possono anche avere interessi concreti

Questo è l'aspetto più brutale, quando anche l'interesse materiale può portare a dire: «Insomma, è anziano, è malato, ha vissuto tanti anni: ora che cosa dobbiamo fare?».

Quindi ciò che ha detto il senatore Romano è fondamentale come il suo emendamento, ma tanto lo respingerete, già lo so. Si sta facendo una legge pazzesca, che consentirà la lite dei familiari intorno al letto. Alcuni lo faranno per un convincimento (perché ci sono persone che hanno una visione diversa), altri potrebbero avere un interesse e noi facciamo una legge che demanda a una pluralità di contesti: pensate ai contenziosi giuridici

quelli indiretti? I figli adottivi, giustamente, sono come i figli naturali, le sorelle, i cugini e fino a quale grado? Gli ascendenti o i discendenti? Chi, in questo contesto? Perché poi si aprirà in sede giudiziaria al primo al primo caso di contestazione di un figlio, di un fratello o di un genitore che contesterà una decisione presa da altri, una discussione pazzesca, anche con profili di ordine penale, perché in questa legge avete scritto un'altra bestialità: e cioè che il medico è esente da responsabilità civili e penali e l'avete scritto perché sapete che si va contro la deontologia medica, prima richiamata dalla senatrice Rizzotti. Quindi il medico viene esposto a delle conseguenze da cui non si salverà con questa menzione, che sarà travolta dalle interpretazioni giudiziarie. Ebbene, l'assemblea dei familiari che cosa deciderà? È un errore gravissimo che deve essere corretto. Non guardate solo l'orologio,

perché ci deve essere qualcosa di ufficiale, qualcosa di concreto, atteso che oggi una persona di mia fiducia può essere mia sorella, domani il mio vicino di casa, dopodomani il senatore Candiani e tra una settimana la mia morosa. La persona deve essere espressamente delegata. Non siamo la *pro loco*, ma il Parlamento della Repubblica italiana: facciamo le cose con criterio, non di fretta. Le cose fatte di fretta producono errori e questo è a sua volta un grandissimo errore.

espressamente delegata a questo. È chiaro che, per come si stanno svolgendo questa discussione sugli emendamenti, le dichiarazioni di voto e queste votazioni, come peraltro è stato enunciato fin da quando in Commissione si discuteva di questa legge, non c'è assolutamente la volontà, ancora una volta, di dare al Paese una buona legge che metta al riparo dalle interpretazioni giudiziarie e mi sembra che i nostri tribunali stiamo facendo semplicemente degli appunti sul disegno di legge, che tecnicamente è scritto malissimo, non si stanno facendo disquisizioni sull'etica o sulla disponibilità o indisponibilità della propria vita:

la circostanza dell'adulto che perde la capacità d'intendere e di volere e che precedentemente definisce come comportarsi. Vi è tuttavia una questione che viene sempre trascurata e che mi angoscia particolarmente: quella del minore.

che lo Stato decidesse chi dovesse vivere e chi non dovesse vivere. Su queste cose bisogna che ci sia una seria riflessione e lo dico con grande dispiacere, perché è una riflessione che scivola via come acqua sul marmo.

Ragioniamo e ragionate, vi prego, su questa eventualità. Qui dentro devono essere messi vincoli seri, severi e molto stretti, perché si sta parlando del diritto di vivere o morire riguardo a persone che non hanno la capacità, nel caso specifico i minori.

vengano riportate in un documento sottoscritto dal medico e dal paziente stesso o da una persona da lui delegata in modo che non ci siano dubbi su quanto sta accadendo. In questo caso praticamente si può

pratiche mediche non consone. Di conseguenza, nel momento in cui un medico pratica l'eutanasia, lo deve scrivere.

non c'è: bisogna solo far sbarrare la casella «la Repubblica», come ha detto prima la senatrice Rizzotti, con la voce «Fatto!». Fate così, ma state facendo uno scempio di fatti poi, quei giornali che vi danno gli ordini, vendono sempre meno copie, perché alla fine parlano di cose che non riguardano la coscienza vera del Paese.

il consenso informato non sia richiesto quando ci si trova in una situazione di emergenza. Questo vale oggi, ma perché non ci sono le dichiarazioni previste dalla norma che stiamo discutendo. Nel momento in cui ci saranno, bisogna evitare che i medici, che devono pensare soprattutto a salvare le vite e la qualità della vita, debbano preoccuparsi della possibilità che il paziente

lo stesso motivo espresso dal senatore Malan ritengo che, in caso di emergenze e di rischio, il medico debba essere libero di poter operare nel migliore dei modi.

al termine «condizioni» di un paziente che sottoscrive il consenso informato. Sappiamo che molto spesso i pazienti non vogliono essere informati o non sono in grado di comprendere, se non in termini molto semplici, quello che può essere un percorso terapeutico, a maggior ragione se hanno un livello culturale non appropriato a comprendere tali informazioni. Anche a proposito del consenso informato, vorrei ricordare un piccolo particolare fondamentale del il consenso informato è un atto stipulato e firmato da una persona in grado di intendere e volere nel momento in cui si presenta una situazione di patologia per per cui ricorre alle cure del medico di una struttura ospedaliera. È quindi attuale al momento in cui il paziente lo deve firmare. Le disposizioni anticipate di trattamento, invece, sono un atto che precede, magari di decenni, una situazione nella quale la persona si troverà. Ora, penso che, anche per poter avere un'uniformità e un testo che sia in grado di essere recepito, qualsiasi sia il livello culturale della persona che lo firma,

Grazie Grazie

«è documentato», le seguenti parole: «salvo che per prestazioni sanitarie implicanti rischi minimi». Ne verrebbe, di conseguenza, che se noi accentuiamo ancor di più questa contrattualizzazione, sarà sempre un rapporto ad incidere e a perdersi nell'ambito della relazione di cura. Se cioè noi accentuiamo sempre più la contrattualizzazione - lasciate che usi questa espressione - il paziente e il medico non saranno mai amici morali, anche per quanto riguarda

Io lo ringrazio per la sua disponibilità rilevando, nel contempo, che qui si riconosce la necessità di migliorare questo testo e che accettare la conversione in ordine del giorno del suo emendamento è un atto di buona volontà del senatore Romano per evitare l'automatismo soppressivo di voti contrari. Tuttavia, rilevo che l'ordine del giorno accolto dal Governo denota che ci si rende conto del fatto che su aspetti che sembrano di dettaglio,

il mio emendamento è volto a specificare, espressamente a tutela del paziente, chi può prestare il consenso informato per suo conto, quando questi non sia in grado di comunicarlo.

chi deve dare il consenso informato, nel caso in cui i familiari non abbiano ricevuto l'informazione, è questo il momento di dire stiamo disciplinando chi esprime il consenso e la forma del consenso. Tenuto conto di quanto abbiamo scritto al comma 3, è evidente che va disciplinato chi deve esprimere il consenso ove il paziente non possa farlo e quali forme si devono assumere.

che bisognerà individuare chi è il familiare, l'amico o la persona di fiducia che dovrà esprimere il consenso. Poiché tutto ciò qui non c'è più, più, l'emendamento tende a dare una certezza matematica su chi debba esprimere il consenso ove il paziente non possa farlo, tenuto conto delle notizie già ricevute in base al comma 3. Questa è la situazione. Volete andare avanti, fatelo pure, però mi sembra abbastanza assurdo anche trasformarlo in un ordine del giorno, lascia il tempo che trova. Almeno il Governo si assuma la responsabilità di dire qual è la forma che deve assumere il consenso, nel momento in cui il malato non è in condizione di farlo, e quale dei familiari o la persona di fiducia che ha ricevuto l'informazione deve esprimerlo. Questa è una questione abbastanza chiara che va risolta, altrimenti è come se non avessimo fatto una norma,

Grazie Il ruolo e il significato del consenso o del dissenso alla cura non deve infatti essere visto come il fondamento dell'attività medica, bensì come il suo limite. L'attività medica intanto è legittima e doverosa in quanto sia diretta al bene integrale della persona cioè alla salvaguardia della sua vita e della sua integrità psicofisica, nonché alla cura e all'alleviamento della sua sofferenza. Il consenso al trattamento non è qualcosa che si può contrapporre al principio di beneficialità, bensì è la partecipazione consapevole del malato alla realizzazione del proprio bene.

psicologica profonda e depressione proprio in virtù di una patologia. Questo aspetto l'avevamo già sottolineato nella legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative,

crea una fortissima depressione, una paura di vivere della persona che ha subìto un infarto. La stessa cosa succede molto spesso con i paziente oncologici, ai quali cerchiamo - pur con le carenze del nostro Servizio sanitario nazionale - di dare un supporto psicologico per poter superare o vivere al meglio

del suo stato emotivo alterato. Ora, credo che tutto ciò debba essere tenuto in considerazione soprattutto per patologie curabili. Questo emendamento vuole riportare alla normalità di una corsia medica, in un rapporto medico-paziente e in un'alleanza terapeutica che in questo disegno di legge vengono totalmente calpestati, questi principi fondamentali.

Signor Presidente, io rispetto tutte le opinioni. Chiedo però ai colleghi di leggere il testo

Che bisogno abbiamo di instillare il sospetto che ci siano medici assassini? Sinceramente mi sembra troppo.

si aggiunge però che il rifiuto non produce alcun effetto quando da esso possa derivare un concreto pericolo di vita non già esistente: una persona che sta bene e che rifiuta un trattamento nel momento in cui non è in condizione di pericolo di vita

si debba tenere conto di questa volontà, perché sarebbe una volontà suicida, autodistruttiva, autolesionistica. Questo è il tema ed è un tema importante, di cui forse lo scadenzario

della situazione; quando invece il rifiuto si è verificato in un momento diverso da quello in cui si trova a intervenire il medico, in cui è è subentrato un concreto pericolo di vita non già esistente al momento del rifiuto, quindi non già programmabile, prevedibile al momento del rifiuto, come deve operare il medico?

che ha fatto un giuramento deve intervenire o avrà dei momenti di esitazione perché abbiamo detto che il rifiuto è valido e non abbiamo escluso la possibilità di invalidare di quel rifiuto ove subentri un concreto pericolo di vita?

di fronte a voi che non dite nulla, il medico non saprà come interpretare il vostro silenzio. Anzi, dal vostro voto contrario capirà che bisogna tener conto del rifiuto, anche in presenza di un concreto pericolo di vita subentrato successivamente, tale per cui non deve intervenire. Questa è la vostra valutazione? Non credo.

garantite in modo artificiale, costituiscono, secondo la dottrina medica, cura e non terapie. Vorrei ricordare che quest'Assemblea pochi anni fa, a larga maggioranza, credo al 90 per cento, affermò ciò. Lo dico in particolare al collega Zanda, che fu firmatario di una mozione, che ho disponibile e che potrei leggere, nella quale il Gruppo del Partito Democratico (prima firmataria la senatrice Finocchiaro e secondo firmatario il senatore Zanda e con loro molti parlamentari) in occasione del cosiddetto caso Englaro ebbero a indicare i criteri di un intervento legislativo in questa materia e tra questi ebbero a sottolineare proprio ciò che ho detto all'inizio del mio intervento e cioè che idratazione e alimentazione non costituiscono terapie, ma cure della persona. È ben vero che anche le cure della persona, che si riferiscono quindi a quella doverosa assistenza umanitaria e ai suoi bisogni vitali, non sono illimitate; è evidente però che a questo proposito devono esistere ragioni molto particolari di appropriatezza dei trattamenti che devono condurre anche a una rinuncia in questo ambito, quando cioè gli effetti possono essere più dannosi dei benefici per la persona stessa.

non assoluta, perché la giustizia creativa vi ha preceduti: la giustizia creativa, in quel caso, arrivò ad inventare perfino un protocollo farmacologico di accompagnamento alla sottrazione di cibo e acqua, ma com'è noto esistono creatori di diritto *legibus soluti* che in quel tempo decisero di agire in questo modo.

Innoveremmo anche rispetto a ciò che pochi anni fa questa Assemblea aveva largamente deciso, certo in un'altra legislatura, verrebbe dire anche con un altro Partito Democratico, con altri gruppi dirigenti di quel partito. Torno sempre su quel punto, che non posso politicamente non rilevare in questa discussione: ho conosciuto un tempo in cui il grande partito della sinistra era più cauto su queste materie e più attento al sentire comune del popolo e ho ho visto via via un'involuzione verso, invece, il luogo comune di alcuni ambienti elitari, a proposito cioè dell'uomo nuovo e dei tanti modi in cui si dovrebbe costruire questo uomo nuovo. Mi viene da chiedere cosa sia successo dal 2009 ad oggi, se il Partito Democratico allora diceva che idratazione e alimentazione non costituiscono terapie e oggi invece vuole codificare con legge che esse sono terapie e come tali rinunciabili, nonostante le gravi sofferenze che, anche in uno stato di sedazione profonda, ragionevolmente comportano per la persona. L'unica cosa che - mi viene da constatare - è cambiata nel Partito Democratico è che il suo gruppo dirigente oggi più di ieri è fatto da cattolici, mi pare di capire molto, molto adulti. Signor Presidente, in effetti ci fu un momento - io c'ero e l'ho vissuto - qualche anno fa, in cui il Senato visse una giornata drammatica, piena di tensione e di emozione e ricordo ancora l'urlo con cui il senatore Quagliariello diede la notizia, mentre parlavamo dello stesso argomento di cui stiamo parlando oggi, della morte di Eluana Englaro espresse anche giudizi pesanti sulle responsabilità che avevano portato a quella morte atroce. Ricordo infatti che siamo partiti da un caso, che si potrà ripetere, di una persona che non era affatto gravemente malata e non soffriva affatto;

amorevolmente curate in istituti che garantiscono la dignità della loro vita anche se hanno delle imperfezioni. So che alcuni colleghi sono nostalgici del tempo,

tutta l'Italia si interrogò. Il Partito Democratico, in quella occasione, sottoscrisse un documento, in accordo con il resto del Parlamento, in cui si diceva che comunque nutrizione e

per provocare una svolta così radicale e per aprire la porta a vicende come quelle che abbiamo vissuto? Torno a riproporre il problema. Penso alle migliaia di persone che sono assistite - bambini, minorenni e piccoli - negli istituti che seguono

Io sono dell'idea che sopprimerli ci riporti alle barbarie del secolo passato. Questo è quello che sta succedendo in Europa e ciò a cui

muore per la patologia che ha, muore sedato senza soffrire, non muore perché viene fatto morire, quindi con un'eutanasia passiva. Questo è un punto fondamentale, su cui richiamo l'attenzione dei colleghi, perché quando, di qui a pochi mesi e anni,

«Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici». Questo è quello che prescrive

non voglio suscitare il nervosismo di nessuno, ma credo che su questo punto sia doveroso poter intervenire con pacatezza e calma, ma anche con quella che, a nostro avviso, è un'oggettiva considerazione dei fatti.

Pregherei però di non mostrare insofferenza, sapendo che si vota domani, se qualcuno in questo dibattito - in cui viene cangurato di tutto e di più - fa considerazioni importanti sul concetto di

un principio fondamentale, considerando in talune circostanze la nutrizione e l'idratazione un trattamento sanitario. È di questo che stiamo parlando. Alcuni di noi non ritengono che ciò sia corretto;

però che sia giusto esporre in quest'Assemblea perplessità sulla definizione della nutrizione e dell'idratazione artificiali quali trattamenti sanitari. Il cibo e l'acqua, infatti, in questo modo vengono parificati a trattamenti medici se assunti attraverso ausili artificiali. Questo è il punto.

l'idratazione e la nutrizione non sono trattamenti sanitari. Non lo dicono i senatori Gasparri, Sacconi o Giovanardi: è un concetto definito nelle regole fondamentali internazionali della scienza medica.

questo che si sta consumando. Ecco perché noi parliamo della deriva eutanasica, ecco perché diciamo che la legge fatta così è un disastro e sarebbe stato meglio affidarsi all'alleanza terapeutica tra famiglia medico e malato.

intervengo soltanto per un minuto. Mi permetto di parlare come medico: ho sentito i colleghi che parlavano di nutrizione e di alimentazione. esame dice che si devono sospendere l'idratazione e l'alimentazione, accompagnando ciò con una sedazione profonda.

che condiziona la sopravvivenza, mentre l'alimentazione serve per far sì che il metabolismo all'interno dell'organismo possa avvenire. La legge

è fisiologica e normale. Questa legge porta alla sospensione dell'idratazione e dell'alimentazione. L'alimentazione non fa altro che assicurare i processi del metabolismo all'interno dell'organismo, perciò quando i colleghi richiamano l'attenzione

credo che dovremmo prendere in prestito una locuzione usata dal senatore Romano: almeno qui dentro, siamo amici morali.

come se tutto potesse ridursi alla rappresentazione di persone che non aspettano altro che ammazzarsi e suicidarsi e di professionisti e familiari che non aspettano altro che spegnere vite in bilico: non è proprio così.

delle storie, che sono fatte di donne e uomini, che si incontrano e devono prendere decisioni complicate e che in questo investono ciò che hanno vissuto e ciò che pensano ancora di poter vivere dignitosamente: di qui il concetto di legge mite. In qualche passaggio e in qualche emendamento, che per fortuna è stato respinto, non ho visto questa idea di legge mite, ma l'idea di una normazione molto rigida, quasi una specie di sollecitazione a cure di Stato a cure di Stato! - e ciò non va bene e non è quello che credo, anche sulla base del mio vissuto professionale, le persone desiderino. Sulla storia della nutrizione e dell'idratazione artificiali,

più volte citati in questo dibattito. Proprio nell'ultimo codice del 2014 arrivammo all'individuazione della tematica nutrizione e idratazione,

Ripeto, in alcuni contesti sono strumenti salva vita nel vero senso della parola. Pensate ai bambini che nascono con la sindrome dell'intestino corto e non hanno altra speranza che un trapianto di intestino: sopravvivono grazie a nutrizione e idratazione artificiali, nell'attesa di un trapianto che che possa risolvere il problema. Pensate a grossi interventi chirurgici, soprattutto sull'apparato digerente e non solo, che nei primi venti-trenta giorni possono solo essere supportati da una terapia totalmente sostitutiva della nutrizione. Quindi, stiamo parlando di presidi sanitari a tutti gli effetti.

Non esistono cure senza terapie; non si può soltanto alleviare la persona senza offrirgli uno strumento ragionevole e consolidato di miglioramento, di guarigione. Questi sono gli scopi della moderna medicina: spesso guarire, ma sempre prendersi cura. Sono distinzioni vecchie quelle tra terapia e cura.

Non ero in Senato, ma affermava una cosa giustissima, così come - fate attenzione, mi rivolgo al senatore Caliendo - la sentenza della Cassazione che rinviò al tribunale d'appello il caso Englaro. Già in quella sentenza c'era scritto che a nessuno può essere consentito di sospendere nutrizione e idratazione artificiali,

che a nessuno, per scelta terza, può essere consentita la sospensione, ma è un trattamento su cui intervengono solo due casi: il primo, che vada a costituire accanimento terapeutico; il secondo, quando interviene una volontà

Senatore Giovanardi, credo che questo provvedimento possa anche evitare che qualche altro tribunale decida come nel caso Englaro. La stiamo facendo o no per questo?

Signor Presidente, entriamo in uno dei temi più conflittuali di questo disegno di legge. Io vorrei usare una argomentazione razionale, sostanziale, non formale né strumentale.

Nell'ambito del biodiritto non esiste una legge mite. Esiste solo una legge giusta. Non è l'aggettivazione della mitezza della legge che rende la legge per sé accettabile, ma la legge si richiama ad un principio di giustizia; e c'è un solo aggettivo che si può abbinare alla legge, che è quello, appunto, della legge giusta. L'amicizia morale, come diceva Engelhardt, non è una semplice condivisione formale ma è la condivisione sostanziale alla luce di principi e valori di riferimento che si condividono. Questa è l'amicizia morale.

Ma è quello stesso codice deontologico che richiama in maniera inequivocabile il ricorso alle dichiarazioni e non alle disposizioni. Quindi, il codice deontologico, se vogliamo richiamarlo, richiamiamolo tutto. Voglio, però, entrare immediatamente nel cuore di questo tema, che è delicatissimo, in cui si esprime in una maniera forte (cosa per me del tutto originale) che una legge definisca cosa, in ambito biomedico, è un trattamento e cosa non lo è. per un motivo molto semplice: qualsiasi cosa in medicina è frutto di una convenzione; è frutto di uno stato dell'attività di ricerca assistenziale che fa classificare il ricorso a un trattamento se sia un trattamento terapeutico o un trattamento di cura. di cura. Ne consegue che se si usa questa terminologia e si dice che «Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale», io sottopongo alla vostra attenzione questa riflessione: ogni legge che specifichi qualcosa esclude altro. Per una sorta di deduttivismo logico io devo trarre questa conclusione: se, solo e soltanto perché la legge richiama esclusivamente nutrizione e idratazione, sono trattamenti sanitari, io devo ritenere che la ventilazione artificiale non è un trattamento sanitario. Mi sarei infatti aspettato, all'interno di questo comma, l'introduzione in questa logica anche della ventilazione artificiale. Quindi, chi approverà questo emendamento sappia che va a ratificare che la ventilazione artificiale non è un trattamento sanitario ma è un sostegno vitale. Una ulteriore osservazione vorrei porre alla vostra attenzione. Non è il ricorso a una prescrizione medica o l'intervento del personale sanitario che tipizza il trattamento come sanitario. Noi usiamo erroneamente una sinonimia tra trattamento sanitario e trattamento terapeutico: non è assolutamente così. Basta un banalissimo esempio: le cure palliative e le terapie del dolore, che sappiamo tutti essere di intrinseca eticità che ne dà luogo alla condivisione, richiedono l'intervento di personale sanitario altamente specializzato. Le cure palliative e le terapie del dolore richiedono l'intervento di prodotti elaborati da case farmaceutiche o da laboratori, con l'intervento con l'intervento dei medici. Mi dovete spiegare, allora, delle due, l'una: o le cure palliative e le terapie del dolore sono trattamenti, anche questi sanitari, intesi come terapeutici, oppure non lo possono essere, perché non svolgono un'azione terapeutica. È vero che la cura contempla la terapia - argomento, questo, a me molto caro - ma non si può esaurire nella terapia; la terapia, infatti, è finalizzata alla guarigione di una persona, mentre la cura è finalizzata non più alla guaribilità di una persona, ma all'assistenza della persona laddove questa è inguaribile.

vuoi che lo definiamo sanitario, vuoi che lo definiamo terapeutico, vuoi che lo definiamo di cura), modalità di nutrizione o idratazione artificiali tutt'ora efficaci, debbano essere considerati trattamenti sanitari». Credo che questo emendamento ricollochi in un perimetro di correttezza clinica, relazionale ed etica la nutrizione e l'idratazione. Detto in altri termini, laddove la nutrizione e l'idratazione non hanno più alcuna finalità, c'è tutta la liceità di poterle sospendere. Ma quando? Solamente in caso di imminenza di morte. Se volete, poi, c'è un secondo emendamento, che chiedo alla Presidenza cortesemente di poter illustrare

questa è una dimensione squisitamente razionale, argomentata, assolutamente non condizionata da fattori di pregiudizio e di preconcetto. È nell'interesse del paziente poter dar luogo a un trattamento che, solamente nella proporzionalità,

e spesso il ruolo suppletivo della giustizia ha creato più confusione che altro. Anche nel caso che tanto fece discutere in quest'Aula e fuori, le sentenze della Cassazione non furono poi così chiare.

affermiamo un principio e poi andremo oltre. Piantiamo una bandierina: si fa questa legge, un domani vedremo se andare oltre, come si è fatto per altri temi.

caso c'è un modo confuso di fare la legge che, secondo me, non è casuale da parte di alcuni. I familiari o il familiare sembra una banalità, ma non lo è. Qua c'è una proposta di alleanza terapeutica tra il paziente e il medico in una certa fase, giunti alla fine della vita. Più volte, in queste discussioni, ho evocato un'esperienza che tanti di noi hanno avuto. A me è capitato di assistere persone; poi arriva un momento in cui il medico, o lo stesso paziente, capisce che le forze vengono meno e, quindi, andare oltre sarebbe accanimento terapeutico, che noi abbiamo proposto di vietare in maniera più più esplicita, ma avete detto «no» pure a quello. Dite «no» se si parla di medico e paziente, dite no se è un familiare perché devono essere i familiari a decidere. Dite no se noi diciamo no all'accanimento terapeutico perché noi accettiamo anche la morte come esito finale.

Condividiamo l'emendamento del senatore Romano e lo voteremo favorevolmente. Il senatore Romano svolge alcune considerazioni non molto dissimili da quelle del collega Bianco, a ben ascoltarlo.

Però, il collega Bianco, al di là del tono, mi è parso sottolineare come la cura della persona costituisca una premessa importante per l'efficacia delle terapie. L'enfasi che ha posto sulla cura e sul benessere della persona mi è parso un motivo in più per garantire per garantire cure; anzi, egli ha concorso a sottolineare la distinzione tra cure e terapie, quella distinzione di cui ha parlato poco fa il collega Romano. Le terapie sono rivolte a curare la malattia e le cure - lo dico atecnicamente - sono rivolte all'assistenza che rivolgiamo alla persona nei suoi bisogni vitali. Non ho compreso come proprio la considerazione sull'importanza delle cure possa condurre a una sorta di equazione per cui, proprio perché importanti, sono rinunciabili tanto quanto le terapie.

che affermava un principio di questo tipo. Il suo punto 11 diceva: «l'idratazione e l'alimentazione, indicate nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente - anche in modo artificiale in quanto fisiologicamente finalizzate al sostegno vitale, non sono assimilate all'accanimento terapeutico e sono comunque e sempre garantite al paziente fino alla fine della vita». Rispetto a questa affermazione si ammette poi un'eccezione un'eccezione che - il collega Romano penso possa convenire - dovrebbe essere nel segno di quel principio di appropriatezza, che dovrebbe presiedere a qualsiasi trattamento, e che egli intende peraltro rinunciabile dal paziente, d'intesa con il suo medico (torna l'alleanza terapeutica), nel momento attuale e concreto in cui si realizza quella volontà, cioè non in modo predeterminato, ma in modo attuale in una situazione di prossimità alla conclusione del ciclo vitale.

l'alimentazione artificiale è sostitutiva di un'alimentazione che potrebbe effettuarsi direttamente ancorché faticosamente, perché esiste deglutizione in molti casi, quindi è un modo di garantire maggiore comodità a coloro che assistono e alla stessa persona che viene assistita. Ma in via teorica e e anche pratica sarebbe possibile un'alimentazione diretta, in due o tre ore circa, probabilmente, rispetto ai *device* impiegati per l'alimentazione artificiale. Ci risiamo. Come non vedere questa ancor più come una zona grigia? Come non vedere ancor più in questo caso la necessità dell'alleanza terapeutica? Come non vedere ancor più in questo caso il bisogno di un'attenzione, di un'affermazione del principio rispetto al quale poi possano esservi anche deroghe affidate non ad una rigida norma, ma al concorso di volontà del paziente e del medico?

più volte adottato questo criterio di affermare un principio e di consentirne alcune limitate deroghe. In ogni caso - mi dispiace senatore Bianco, lei sa che la stimo come stimo la presidente De Biasi - non credo sia un buon modo di legiferare quello di inseguire la magistratura creativa. creativa. Noi non siamo qui riuniti per dare ragione al magistrato, che ci ha anticipato con sentenze che dovrebbero, al di là dell'opinione di ciascuno, trovarci uniti nell'affermare il primato del Parlamento e del popolo. Tuttavia, vedo che ormai molti sono acquiescenti ad altri primati che sconvolgono il nostro equilibrio costituzionale.

I dubbi che vengono posti sono assolutamente fondati e legittimi, soprattutto perché si va troppo semplicisticamente a definire ciò che è alimentazione e ciò che invece è cura.

un caro, un congiunto o un amico in una circostanza terminale. Ci sono scelte di volontà, ma anche doveri che si devono rispettare riguardo alla cura della malattia e soprattutto al fatto di dare una risposta che deve essere di vita e non di morte alla fine di un percorso, ma sempre con una prospettiva positiva. Si tratta non di decidere se chiudere o no un percorso, ma di ricordarsi che quando si fanno queste norme si deve legiferare non sul fine vita, ma sul diritto alla vita, che è un principio positivo. Se si invertono i rapporti, si innesca un meccanismo da cui rischiamo di non uscire o, peggio, di uscire

Probabilmente pochi in quest'Aula - o forse sarò stata l'unica - hanno frequentato reparti di terapia intensiva quando autonomamente, in base alla situazione clinica della persona,

In alcuni casi in cui la situazione clinica del paziente lo richiede, già normalmente si sospende l'idratazione perché si creano, negli squilibri dell'organismo, degli edemi importanti che creano dolore e sofferenza, come può essere un edema cardiaco o polmonare. A maggior ragione, magari, si aumenta la quota proteica proprio per far tornare lo squilibrio elettrolitico, in modo da far riassorbire gli edemi.

Mi ha stupito vedere a livello mediatico i casi drammatici e le fotografie dei casi Welby o del dj. Vorrei però ricordare che alle persone capaci d'intendere e di volere la legge già permette di rifiutare le terapie e le cure.

siffatti casi sono stati amplificati per arrivare a questo. È chiaro che togliere la nutrizione e l'idratazione a una persona è un segno di eutanasia mascherata, di cui il medico

stiamo esaminando un disegno di legge, a mia prima firma, per prevenire i disturbi del comportamento alimentare,

anni. Sappiamo perfettamente che togliere nutrizione e idratazione - più idratazione, direi, che nutrizione - porta la persona a morte certa. Quindi, perché non dire che questa è una forma velata di eutanasia? È la realtà. Si abbia il coraggio di dire che, quando una persona rifiuta le cure,

Signor Presidente, chiediamo che, in caso di rifiuto di idratazione e nutrizione, il medico debba accertarsi che il paziente abbia pienamente compreso che la sospensione causerà inevitabilmente la sua morte. Deve esserne

si torna con questi emendamenti sul rapporto tra cure e terapie. Proprio in quanto diverse, è importante che ci sia una specifica informazione almeno nei confronti del paziente, perché la sospensione di idratazione e alimentazione potrebbe rendere meno agevole la stessa somministrazione di cure palliative e di sedazione del dolore. Si può quindi

minore ricettività da parte del paziente ed è bene che di questo egli sia consapevole. In sostanza, ciò di cui stiamo parlando non è affatto un accompagnamento dolce a morte, ma con ogni probabilità è un accompagnamento molto doloroso, che deriva dalla privazione di cibo e di acqua e dalla ineffettività

a seconda che la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico sia o meno cominciata e, quindi, il trattamento sia già iniziato o no sotto la responsabilità medica. caso, cerchiamo di regolare, in quella zona grigia, almeno alcuni presidi riferiti al benessere della persona.

Grazie, l'accertamento volta per volta della capacità di intendere e volere della persona nei casi dubbi, con particolare riferimento al suo stato confusionale, anche temporaneo, o di depressione o di psicosi.

Anche noi vogliamo evidenziare il fatto che la capacità di intendere e di volere debba essere accertata di volta in volta, nei casi dubbi, con riferimento alla condizione di stato confusionale temporaneo o di depressione o di psicosi. Anche in questo caso, quindi, occorrono ulteriori analisi e accertamenti sullo stato del paziente.

noi sappiamo che le buone pratiche cliniche e le linee guida rappresentano un faro, un punto di riferimento. E mi sembra che il comma 6 sia in perfetta sintonia, salvo verificare, però,

Se c'è una relazione di cura, il medico non può rispettare in maniera assoluta, ma deve prendere in considerazione e, insieme al paziente, fare un percorso terapeutico e di cura che sia nell'assoluto interesse del paziente stesso. Voglio portare un esempio di una banalità estrema, per rendere più chiaro questo mio concetto e essere io più chiaro. Se io, profano di architettura, mi rivolgo, non a caso, a un *archistar*, cui dico di voler costruire un *auditorium*

Detto in altri termini e fuor di metafora, se ci sono e riconosciamo tutti una relazione e un'alleanza di cura, il medico deve prendere in considerazione e non può

con il codice deontologico, con la Convenzione di Oviedo, vari altri documenti e i dettami del Comitato nazionale per la bioetica, che - appunto - parla di una presa in considerazione, ma non della imperatività dell'atto stesso.

Il senatore Romano ha descritto - a mio avviso - in modo molto efficace, l'alleanza terapeutica, il dialogo tra il medico e il paziente, o tra il medico, il paziente e i familiari del paziente stesso. Il limite naturale nel carattere vincolante della dichiarazione è intimamente connesso alla scienza e soprattutto alla coscienza del medico. Questo mi conduce, quindi, a considerare molto correlati il tema del carattere non vincolante della dichiarazione e l'obiezione di coscienza, qualora il carattere vincolante volesse essere mantenuto. infatti l'istituto dell'obiezione di coscienza - per fortuna lo rispettiamo - ed è paradossale che in questo provvedimento, di fronte a

Voglio essere molto chiaro a proposito di un aspetto. La senatrice De Biasi in Commissione mi ha sentito dire esplicitamente che non sono qui a proporvi l'obiezione di coscienza delle strutture. Mi dispiace, ma non riconosco coscienza alle strutture: riconosco coscienza alle persone in qualunque struttura esse operino, che sia una struttura pubblica, privata, privata classificata; alle persone sì. Non possiamo contemporaneamente imporre il carattere vincolante delle dichiarazioni e l'obbligo di aderirvi da parte del medico, pena quella responsabilità civile che ormai è sempre dietro l'angolo di una corsia o di una porta d'ospedale, ben al di là della tutela dei pazienti, spesso frequentemente con modalità temerarie. Voglio sempre ricordare che, quando assumiamo la decisione di una norma, quando decidiamo un provvedimento, dobbiamo sempre pensare all'immanente anomalia consistente È un'anomalia che c'è, che abbiamo il dovere di risolvere, che in questa legislatura abbiamo probabilmente aggravato, ma che deve essere sempre chiave di lettura dei nostri provvedimenti nel momento in cui non l'abbiamo ancora risolta.

che non è però quello che dobbiamo riportare in una legge. Dobbiamo discutere tra noi medici, a livello di convegni e congressi scientifici, ma nella legge non possiamo portare la nostra cultura medica. E ricordo, colleghi, che, antropologicamente, la prima terapia è stata l'alimentazione, considerata una terapia fin dall'inizio della vita del genere umano.

autodepurarsi, ha scoperto che il digiuno è la miglior medicina per difendere le cellule dall'aggressione di fattori esterni. Quindi ci sarebbe da disquisire in maniera continua

Dunque, la perfezione che andiamo a cercare porta al massimo dell'ingiustizia. consapevoli della scelta che abbiamo fatto di approvare una legge sul fine vita e sulle dichiarazioni anticipate di trattamento: pur con tutte le imperfezioni, è una legge che vogliamo abbia anche il nostro Paese e, quindi, cercando la perfezione

un comma e non è possibile sostituire il comma di una legge con un ordine del giorno.

Signor Presidente, in questo caso viene valutata, come in altri emendamenti, l'obiezione di coscienza o la convinzione del medico di salvare il paziente.

Grazie di una legge confusa, contraddittoria, per tutte le ragioni che stanno emergendo nell'odierna discussione e che sono chiarissime a tutti, anche a chi respinge tutto.

modificabilità da interpreti plurimi, i familiari di cui sopra, espongono veramente non all'eutanasia ma all'omicidio di Stato. L'emendamento in esame è un'occasione per correggere un errore palese.

vorrei sottolineare la rilevanza di questo emendamento che riguarda il caso della controversia tra il fiduciario e il medico curante.

Vorremmo che questa controversia non venisse risolta in una algida o ideologica aula giudiziaria, ma venisse rimessa a un collegio

Presidente, prima d'intervenire su questo emendamento - e quanto dico è inerente al contesto della discussione - faccio una riflessione dal punto di vista politico, che è la

duemila emendamenti. Io faccio la domanda a me stesso, a tutti coloro i quali sono presenti qui dentro e a tutti coloro che gridano allo scandalo quando si parla di certi argomenti in quest'Aula e una parte della maggioranza non risponde o fa orecchie da mercante.

trovi in una situazione di urgenza sia nell'intubare un paziente sia nel mettere un defibrillatore non può sapere se il paziente ha rilasciato disposizioni anticipate. A questo punto, il medico che cosa fa? Se interviene e gli salva la vita, il paziente lo ringrazia oppure, se interviene e gli salva la vita nonostante le sue disposizioni e il paziente ha delle sequele, questi lo denuncia. Se, nel dubbio, visto che vi sarà anche un problema assicurativo in tutto questo, il medico non interverrà, potrà essere denunciato dai familiari e dal paziente stesso per omissione di soccorso. A questo punto, cosa deve fare un medico in un Pronto soccorso? Ricordiamoci che in quel Pronto soccorso potrà essere ricoverato anche il figlio di qualcuno che siede in quest'Aula e che voterà questa legge, senza possibilità di curarlo.

i medici, dopo che è stata determinata la morte clinica di un infartuato, tentano per altri venti minuti di rianimarlo e molte volte, dopo venti minuti, mezz'ora, riescono a rianimarlo e a riportarlo a una vita di relazione completa: quello non è accanimento. Ma in molti Pronto soccorso questi medici vengono criticati. Infatti, nel momento in cui infartuato appare morto e il cuore non batte più, si chiude la pratica in maniera sbrigativa. Io, invece, sono per una cultura che non chiuda la pratica in maniera sbrigativa.

(che sarebbe un eroe della lotta contro la mafia) sottoscritta da giuristi e medici e indirizzata a tutti i deputati e i senatori questa mattina, a fior fior di professionisti che ci hanno segnalato queste criticità. Se voi pensate di superarle urlando, non le superate. Abbiamo sentito l'ex Presidente di Scienza e vita dirci delle cose assolutamente sagge e documentate (e sono state tutte respinte). Stiamo parlando di cose serie, compreso il comportamento nei Pronto soccorso - e lo vedremo anche negli articoli successivi - nel rapporto tra medico e

Questi sono nodi reali, non solo per chi darà le disposizioni, ma anche per milioni di italiani, che dovranno confrontarsi con questo nuovo clima culturale e con questa nuova accezione di delegittimazione di delegittimazione dei medici. Non risolvete il problema urlando e neanche umiliando il Senato. Infatti, se fossimo in situazioni normali e non in uno *spot* pre-elettorale (che vi ha sempre portato sfortuna: mi ricordo quello sul Titolo V: vi ringrazio perché lavorate per il centrodestra, anche dimostrando questo tipo di chiusura assoluta), se fossimo in condizioni normali di dialettica parlamentare, alcune delle osservazioni fatte dal senatore Romano sarebbero state accettate e, davanti a obiezioni come quelle che sono state mosse dalla collega Rizzotti, ci sarebbe stata attenzione. Ma voi marciate con le urla e non con i ragionamenti. Questi problemi si apriranno tutti. Speriamo che nella prossima legislatura ci sia qualcuno più saggio di voi, come per il Titolo V, che sappia rimediare ai vostri errori.

Presidente, ci sono due esigenze: una secondaria, che è quella di usare la lingua italiana in una legge italiana, così si evita di dover andare a cercare caratteri sulla tastiera e una più importante che

e, quindi, la cosa logica è parlare di «operatori sanitari coinvolti»; anziché tirar fuori una parola un po' vacua che non si sa dove finisce. Coloro che sono coinvolti devono partecipare a questa informazione; quelli che non sono coinvolti no. Sembrerebbe una cosa ovvia.

con questi emendamenti, tra cui quello che, insieme alla collega Rizzotti e altri colleghi del Gruppo di Forza Italia, abbiamo firmato - ma ce ne sono altri analoghi di altri colleghi - chiediamo la soppressione del comma 9 dell'articolo 1, che è fondamentale. In esso

alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti. Noi siamo un Paese pluralista. Esistono strutture sanitarie

strutture sanitarie di vario orientamento. Poi capisco che se uno ha delle convinzioni deve anche tenere conto delle leggi dello Stato ma, al di là che questo provvedimento non consente nemmeno l'obiezione di coscienza al medico, si rafforza la protervia giacobina dello Stato. Quindi, è una legge iperstatalista0 (stavo dicendo «iperstalinista», ma sarebbe un anagramma), la quale legge dice che ogni struttura sanitaria pubblica o privata deve applicare questa cosa complicata. Sposetti, perché? Ci saranno pure le cliniche sovietiche, forse, che non la volevano applicare; non so, guarda nella fondazione se ne hai qualcuna. C'era anche Spallone, che faceva ben altre cose come

queste norme. Noi abbiamo un Paese plurale dove esistono strutture che potrebbero anche rinunciare a convenzioni. Adesso c'è anche tanta immigrazione, quindi prima o poi ci saranno anche gli ospedali islamici, chi lo sa? Come c'è l'ospedale cattolico e quello israelitico, quindi perché escluderlo? quindi che sia necessario eliminare il comma 9 per eliminare questo obbligo illegale, incostituzionale, liberale, vergognoso.

Presidente, come siamo per l'obiezione di coscienza per il medico, siamo per l'obiezione di coscienza per la struttura, per le stesse motivazioni menzionate dal senatore Gasparri. Noi riteniamo che ci siano delle strutture ospedaliere che hanno una *mission* e un codice etico; di conseguenza, non si può pensare di stravolgere quelle strutture ospedaliere. Visto che c'è una pluralità pluralità di strutture ospedaliere, nel momento in cui un malato non vuole avere a che fare con questo tipo di strutture, va in altre e non ci sono problemi. Però a quelle strutture bisogna lasciare la libertà di scelta.

la seduta è ripresa.

sanitari, si può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

o è un atto di irreversibilità, oppure è un dato - *hic et nunc*, qui e ora - che può trovare in un trattamento antalgico o antidolorifico la sua soluzione. Ciò vuol dire anche che se noi estendiamo il termine «sofferenze» ad altri tipi di patologie, come quelle di ordine psichiatrico, si andrebbe a giustificare il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua anche in situazioni di sofferenze di ordine psichiatrico. Infatti,

1 stabilisce che «Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico». il paziente, rifiutando la proposta del medico di alleviare le sue sofferenze con la terapia del dolore, rifiuti ogni tipo di terapia, come già stato detto, a cominciare dall'idratazione e dalla nutrizione. In questo caso, invece, il medico deve deve adoperarsi comunque, indipendentemente dalla volontà del paziente? Mi sembra tutto molto strano.

che si vorrebbe accompagnare con sedazione palliativa profonda e continua, cioè con quel modo di conduzione a morte che abbiamo già conosciuto in un noto caso. Mi sembra che questa sia, ancora una volta, un'espressione che conferma

Presidente, per chi non avesse il testo davanti, l'emendamento prevede che «Il consenso informato, quando incide sulla qualità della vita successiva è espresso dal minore che ha compiuto 16 anni.».

oggetto di interventi che potevano incidere sulla successiva qualità della vita -faccio un esempio: il taglio di una gamba, delle due gambe, la perdita delle braccia - per ragioni cliniche.

Qualcuno sostiene sia necessario tener conto anche della posizione del minore che abbia compiuto gli anni quattordici sotto il profilo del dissenso. Io mi sono limitato alla cosa più evidente: siano i genitori o altri, vi rendete conto che noi incidiamo sulla qualità della vita di un minore che ha già compiuto gli anni sedici? Non mi venite a dire che questa norma deve essere approvata così com'è perché non può andare alla Camera. Vi rendete conto che state facendo una cosa di una gravità inaudita? Poi mi parlate di minori, di tutela dei minori, di leggi che non vengono approvate per la tutela dei minori o di ricerche biologiche: quando un minore ha compiuto sedici anni ha tutto il diritto di poter esprimere il proprio consenso quando può essere attinto da un tipo di intervento che incide sulla qualità della sua vita successiva.

e nipoti, avendo la possibilità di valutare un principio che è di civiltà giuridica oltre che di civiltà sociale, non può lavarsene le mani

a questo punto faccio un tentativo, ma non so quale possa esserne l'esito. Se la posizione è di una preclusione assoluta perché neanche un ordine del giorno possa essere preso in considerazione, ne prenderò atto. Ripropongo, nell'ambito dell'emendamento 3.126, la richiesta di trasformazione dello stesso in ordine del giorno, se tecnicamente possibile, dove si riporta che «Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile

Signor Presidente, questo emendamento, come il successivo, tratta di consenso informato e dei minorenni, su cui si è esercitato poco fa anche il collega Caliendo. Esso stabilisce che i genitori o il tutore esercitano la patria potestà, avendo come scopo esclusivo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore. molto importante, perché questo disegno di legge riguarda soprattutto due categorie di malati: da una parte, quelli che sono colpiti da malattie degenerative e, dall'altra, quelli che subiscono traumi in conseguenza di incidenti. Se lei, signor Presidente, e i colleghi di vedere la letteratura specializzata, vi rendereste conto che in questa seconda categoria rientrano soprattutto giovani, a volte minorenni, a volte che hanno di poco superato la maggiore età. Quello che mi ha colpito è che questi giovani traumatizzati, anche per le loro qualità e capacità fisiche, secondo la letteratura, quando cadono in stato di incoscienza, nel 90 per cento ritornano a svolgere regolarmente le loro funzioni vitali; si riprendono, diciamo con il linguaggio corrente, al cento Lei comprende, signor Presidente, che in una condizione di questo tipo, il tema del consenso informato (e che questo consenso sia dato nell'esclusivo interesse della salute del minore) è molto importante. Questo, infatti, è uno dei punti delicati. Una cattiva informazione potrebbe causare una forte perdita di vite umane, anche di vite che si sarebbero potute del tutto recuperare. Questo, a maggior ragione se è vero quello che dice il collega Caliendo, su cui ho dei dubbi; ma, se è vero che è necessario parere anche di un sedicenne e, in qualche modo, della sua dichiarazione anticipata, è ancora più importante che il consenso informato sia effettivo e che questo sia reso

che fa riferimento agli articoli 23, 24 e 25 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che abbiamo ratificato nel 1991. Questo articolo è maledettamente delicato, proprio perché riguarda giovani e disabili e ricordo un bellissimo intervento della senatrice Bignami, nei giorni scorsi, in sede di discussione generale, a questo proposito. Ci auguriamo che davvero, anche con le preoccupazioni legittime circa la possibile giurisprudenza del giorno dopo, questo non diventi l'articolo della rupe Tarpea,

Grazie,

non già perché non abbiamo il pieno rispetto della dignità del minore che si trovi in questa situazione ma, al contrario, perché questa espressione è estremamente ambigua. Lo abbiamo visto nel caso di Charlie Gard, il bambino

con la bella ragione che poteva essere troppo stressante per questo bambino affrontare il viaggio. L'alternativa era morire.

che questo bambino patisce un viaggio per uscire dall'ospedale: è meglio farlo morire. Questo articolo 3, a mio parere, è quello più importante di tutto il provvedimento, perché riguarda i minori e i minori possono essere sia dei sedicenni o diciassettenni, che sono pienamente in grado di esprimere il proprio parere sulle cure, specialmente se sono in condizioni tali da affrontarle, perché si matura molto rapidamente in quelle circostanze, sia bambini totalmente privi della possibilità, anche se in piena salute, di esprimere qualsivoglia consenso o diniego. Togliere queste parole darebbe quindi un elemento di

devo dire che la richiesta di trasformarlo in ordine del giorno e il rifiuto da parte del Governo di accogliere l'ordine del giorno è molto emblematico, noi potremmo intendere che il Governo e la maggioranza, determinati come sono all'approvazione definitiva di questo testo, votino talora anche contro contenuti di buon senso, che altrimenti si immaginerebbero largamente condivisi. In questo caso, esprimere il parere contrario su un emendamento che chiederebbe di interpretare questo articolo in base alla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia

alla retorica corrente su questo sistema e su tutti i suoi prodotti, però vi sono alcune Convenzioni fondamentali che almeno costituivano, fino a poco tempo fa, un pavimento condiviso, con l'unica eccezione di Paesi in condizioni molto arretrate, soprattutto dal punto di vista istituzionale. Constato che noi stiamo regredendo, stiamo scendendo al di sotto di quel pavimento e la furia eutanasica vuole travolgere anche minori e disabili. *(Proteste dal Gruppo

Signor Presidente, ancorché del tutto superfluo, perché avendo noi ratificato la Convenzione non capisco per quale motivo dobbiamo ripeterlo, chiedo al Governo

PD)*. Per me è superfluo, ma se vogliamo fare un ordine del giorno in cui si rafforza la Convenzione ONU, io personalmente non ho problemi. qualche problema di maliziosità rispetto al fatto che si definiscano solo alcuni articoli; pertanto, se il senatore Sacconi fosse d'accordo a mantenere il richiamo all'intera Convenzione, chiederei al Governo di rivedere la sua posizione.

Come membro della Commissione infanzia posso affermare che abbiamo richiamato molte volte in quest'Aula questa Convenzione, ratificata dal Parlamento italiano. Andare a cercare cavilli, in realtà per non tutelare

in questo caso il parere del Governo sarebbe favorevole all'accoglimento, sempre rimettendosi all'Assemblea. Il parere precedente è stato espresso sulla base del fatto che questo Paese ha sottoscritto quella Convenzione, che non va sempre richiamata, perché se ogni volta richiamassimo le convenzioni sottoscritte, i testi

perché mentre quello trattava del consenso informato al trattamento sanitario del minore, nello specifico l'emendamento 3.126 tratta del consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo

Si ipotizza il conflitto fra il rappresentante dell'incapace che rifiuta le cure proposte e il medico che ritenga invece le cure appropriate e necessarie, rinviando la risoluzione del conflitto al giudice tutelare. Dunque la decisione sul ricorso, proponibile tanto dal rappresentante di chi rifiuta le cure, Grazie, la decisione rispetto a questo conflitto ad un soggetto medicalmente non competente qual è il magistrato; *pardon*, il magistrato è competente su tutto e, com'è noto, ho ricordato che ha anche elaborato protocolli farmacologici originali,

dar luogo quindi ad una composizione che tenga conto di tutti gli elementi che concorrono a definirla.

tra il rappresentante legale o l'amministratore di sostegno di persona interdetta o inabilitata e il medico, che ritenga che le cure siano invece

Oggettivamente la soluzione peggiore è quella di demandare la decisione al tribunale; è probabilmente la più inumana, quella che fuoriesce completamente da quel concetto di alleanza terapeutica che qui viene interpretato in maniera differente, ma che nessuno di noi ha rigettato. In un caso come questo e se il conflitto è di questo tipo, noi riteniamo che la soppressione del del comma 5 consentirebbe di far prevalere il giudizio informato, oggettivamente

nemmeno per cercare di comprendere quali soluzioni possono derivare dall'esperienza di episodi effettivamente accaduti. Per questo motivo, chiedo ai colleghi un attimo di riflessione sull'emendamento 3.5005 e un voto anche simbolicamente maggiore rispetto ai voti che gli emendamenti fin qui discussi hanno raccolto.

nel momento in cui c'è un conflitto tra i legali rappresentanti (ossia i tutori del bambino) e i medici, sono andato a riguardare i commenti dei politici italiani di quei giorni.

che persino Papa Francesco ha scritto un *tweet* (ormai anche il nostro Papa scrive i *tweet*): «difendere la vita umana, soprattutto quando è ferita dalla malattia, è un impegno di amore che Dio affida a ogni uomo.» Signori,

prevedibile si potrà realizzare nelle situazioni in cui non c'è il deposito di una DAT (che adesso non vorrei definire disposizione e preferisco chiamare dichiarazione anticipata di trattamento), o quando si creerà un conflitto tra il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata (o l'amministratore di sostegno) e il medico.

del Comitato etico indipendente, dove sono rappresentate competenze e specializzazioni varie e anche sentieri diversi, che rappresentano un punto di riferimento certo. Si tratta di una sorta di stanza di compensazione, a evitare che la conflittualità si trasferisca nella dimensione contrattualistica e nella giurisdizzazione direttamente in un tribunale. Ecco i motivi per i quali chiedo che già prima di arrivare in sede di tribunale, si possa chiedere il parere, cosa che già avviene oggi e che rientra nelle competenze

genitori? Sicuramente la maggioranza degli italiani la pensa in questa maniera. Il problema è che nella legge al nostro esame viene scritta una cosa totalmente diversa. La leggo perché ci sia chiarezza: il «il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie». È il caso contrario di quelli citati, ma questa logica, dando al tribunale la possibilità di intervenire, si estende a 360 gradi.

per evidenti ragioni non possono esserci per un bambino di due-tre mesi o di un anno o due anni - prevalgono le azioni a maggior tutela della sopravvivenza del paziente. Si opta cioè per la vita, si opta per il medico, si dà la possibilità al medico, dal punto di vista scientifico, metodologico e delle attività che possono salvare il bambino e non si dà prevalenza alla dichiarazione, che invece vuole che il bambino venga soppresso nella maniera che sappiamo, facendo venir meno

il cinismo con cui si sta procedendo, perché non c'è nemmeno una contrapposizione tra una presunta maggioranza e le opposizioni. Il senatore Romano, che appartiene ad un altro schieramento, ha fatto, su un punto del disegno di legge, osservazioni ragionevoli,

va meglio, perché il linguaggio è più consono alla modernità. Potremmo dire che è pro vita, perché dice che in caso di contrasto le ragioni della sopravvivenza devono prevalere.

che porteranno - quelli sì - a contrasti giurisdizionali. Credo quindi che approvare l'emendamento in esame sarebbe un atto ragionevole: non mi faccio illusioni, ma perseveriamo nella buona causa e nelle buone proposte.

il rappresentante legale della persona minore, che rifiuta le cure, e il medico che ritenga invece che le cure siano appropriate. Quando c'è questo conflitto - posto che

interdetta o inabile - si ricorre al giudice tutelare e, come dice il testo della legge «la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria». Quindi, c'è una pluralità di soggetti che può avviare il ricorso rispetto a questo contenzioso. A me pare che ciò costituisca una maggiore tutela

che dovrebbe consentire che si realizzi al meglio l'alleanza terapeutica tra medico e familiare o legale rappresentante delle persone disabili o minori.

Signor Presidente, nel corso della discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità, a proposito di questo provvedimento, ho avuto modo di sviluppare un ragionamento che, a partire da un'idea di antropologia pessimista, intendeva elaborare la categoria di autodeterminazione come principio costitutivo della personalità umana. Avendo ricevuto nel merito alcune garbate critiche, avrei molto volentieri voluto rispondere in questa sede,

Lasciate ai genitori la facoltà di decidere per la vita dei loro figli, non lasciategli altro, perché direi che, nelle condizioni in cui debbano fare queste scelte, i genitori non sono in grado di intendere né tanto meno di volere.

veramente stare i minori, lasciate stare i disabili. Se c'è qualcuno ammalato che vuol mettere fine alla sua esistenza, io non sono in disaccordo. Qui nessuno è in disaccordo.

Romano, chi lo ascolti. Adesso sopprimiamo l'articolo 3 e votiamo tutti insieme questo bel disegno di legge. Vi lascio con il comma 4 3, per dar senso al senso di questo articolo. «Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata».

la parola non solo per annunciare il mio voto contrario all'emendamento che ci accingiamo a votare a scrutinio segreto, ma anche per esprimere in questa sede il mio sincero apprezzamento e sostegno al lavoro dei tanti colleghi che hanno sostenuto e stanno sostenendo l'opportunità di approvare questo disegno di legge. Insieme ai senatori Monti, Rubbia e Piano ho avuto già modo di argomentare pubblicamente l'opportunità e l'urgenza di portare a compimento questa riforma. Questa decisione si può realizzare solo votando contro ogni ipotesi Questa decisione si può realizzare solo votando contro ogni ipotesi emendativa che è stata formulata e in tal senso orienterò tutte le mie scelte di voto

voglio davvero ringraziare tutti i colleghi che stanno scrivendo una importante e non più rinviabile pagina della storia parlamentare di questo Paese. *(Brusio. Richiami del Presidente).* Da cittadina, in questo fine legislatura, voglio esprimervi una gratitudine sincera per

che bisogna avere anche una certa misura. Si può anche non essere presenti ai lavori del Senato, perché è qualcosa che riguarda ciascuno di noi, ma francamente farlo in questo modo, in una finestra di opportunità di presenza, forse è un po' offensivo nei confronti di tanti colleghi che sono stati presenti qui ieri e oggi e che saranno qui domani. *(Applausi

evidentemente non avrebbe, poi, il tempo di essere approvato. Da un punto di vista simbolico, evidenziare quanto è chiaro a tutti

Credo, signor Presidente, con molta sincerità, con la stessa sincerità con la quale mi sono espresso, che se non vi fosse il vincolo di cui sopra, cioè il fatto di non poter correggere il disegno

dissidenti rispetto a questo modo di procedere, che sono stati in quest'Aula ieri e oggi e che ci saranno anche domani. Presidente, voteremo a favore di questo emendamento perché anche questo segue la logica che stiamo proponendo ormai da giorni: non più disposizione, ma dichiarazione. ma dichiarazione. Sembra una stupidaggine la differenza tra dichiarazione e disposizione, ma con la disposizione si obbliga qualcuno e con la dichiarazione no. Presidente, in questo momento con il mio intervento rappresento anche il senatore Volpi, che è uscito dall'Aula. Ricordo sommessamente alla senatrice Cattaneo che i signori Monti,

la definizione di dichiarazione in luogo di disposizione, ma soprattutto, nel caso delicatissimo dei minori e dei disabili, vuole, con la sostituzione del termine, indicare il carattere non vincolante ma di mero orientamento dei contenuti della dichiarazione. [SCILIPOTI

la previsione di un'eventuale futura incapacità non può essere altro che irreversibile perché l'incapacità, sotto il profilo biomedico, può presentare le graduazioni più varie e, di conseguenza, è solo in ragione della irreversibilità ad autodeterminarsi che si può dar luogo all'attuazione della DAT sottoscritta. Questo è il motivo per cui ritengo che l'irreversibilità sia l'elemento caratterizzante. Se non c'è irreversibilità, ne viene di conseguenza che quanto riportato all'interno delle DAT potrebbe essere controproducente *quoad vitam* per il paziente e per la persona che le ha sottoscritte. Quindi voglio dire che queste volontà poi devono essere prese in considerazione sempre nell'ottica di una dichiarazione e non di una disposizione. Mi sembra che questo emendamento risponda a un principio di ragionevolezza; ritenendo che risponda a tale principio, mi farebbe piacere che possa intervenire qualcuno che mi dimostri l'irragionevolezza.

che venga garantito il modo. Già abbiamo appurato questa mattina che avremo per un periodo di tempo venti sedi regionali dove potranno essere depositate queste disposizioni, più una sede nazionale che è

Signor Presidente, questo è un altro dei punti controversi di questo provvedimento che vede in dissenso anche chi, come me, è favorevole a che ci sia una legge sulle dichiarazioni anticipate. L'emendamento riafferma il divieto di sospensione di idratazione e nutrizione artificiale - vorrei un attimo di attenzione - qualora questa comporti la morte del paziente per disidratazione o denutrizione. cioè vietata quando la morte è dovuta a queste cause e non alla patologia del malato, vale a dire quando il malato, a causa della sospensione della nutrizione o della idratazione, muore non per la sua malattia, ma fondamentalmente per la mancanza di idratazione, che chiaramente come morte di quella per la mancanza di nutrizione. Per tale ragione noi chiediamo che in questo caso idratazione e nutrizione non possano essere oggetto di dichiarazioni anticipate di trattamento e quindi rientreremmo nelle dichiarazioni, prendendo distacco da ipotesi eutanasiche. Inoltre, e questa mi sembra un'altra previsione di buon senso, si richiede che l'indicazione di un soggetto fiduciario sia una facoltà

l'istituto del consenso informato e quello delle DAT. Sappiamo benissimo che le DAT, espresse ora per allora, potranno essere libere, ma forse non informate, perché nelle DAT non si contempla la sottoscrizione dell'informazione da parte del medico. Un *vulnus* ulteriore è riportato in questo comma 2, perché si dice che «L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT». Benissimo, perché significa che si è creato un rapporto di fiducia nel riconoscere una persona che rappresenterà lo stesso nelle sue incapacità e inabilità. Ma si aggiunge anche che c'è la possibilità di dare luogo all'accettazione con atto successivo allegato alle DAT. DAT. In italiano cosa vuol significare? Che si sottoscrivono le DAT e si rimanda a un tempo successivo, che non si identifica quale possa essere, l'indicazione e la definizione del fiduciario.

in questo interregno temporale il medico assisterà la persona che ha sottoscritto le DAT nell'ambito delle quali ci saranno delle volontà che potrebbero essere

Deve ricorrere al magistrato, cioè davanti all'emergenza - appunto *ictus*, trauma cranico o infarto - e alla possibilità di salvare il paziente, deve andare ad aprire una controversia dinanzi ad un magistrato. Bella scelta di civiltà. con la valutazione di un collegio di medici, che può immediatamente intervenire o impedire che anche la vita o la morte di una persona in questo Paese siano messe in mano ai vari Ingroia, cioè ai magistrati. Ce ne sono di bravissimi, ma ce sono anche di totalmente incompetenti ad entrare in questioni così delicate. Viene dunque esautorato il medico,

a mio parere - tendenzialmente negativa. Invece, ci si affida a un altro caso, cioè al giudice. Pertanto il pericolo, che è è stato consolidato con l'approvazione dell'articolo 3 riguardante la situazione dei minori e degli incapaci, che si verifichino fenomeni molto simili, sia pur non uguali, al caso di Charlie Gard, c'è. Andiamo così contro quelle bellissime dichiarazioni che praticamente tutte le forze politiche hanno rilasciato all'epoca del terribile avvenimento che ha riguardato Charlie Gard.

prende in considerazione le DAT e le valuta senza sentire il fiduciario. Delle due l'una: o il fiduciario ha un ruolo dialogico e costruttivo in una relazione di cura, oppure Ne viene un'altra conseguenza, perché bisogna prendere in considerazione - non solamente rispettare - le DAT per renderle attuali. Abbiamo sempre detto che le DAT non sono attuali, perché in questo momento, ora, posso decidere per quando sarà - - scaramanticamente posso dire il più tardi possibile - ma evidentemente non potrò fare altro che valutare in maniera generica le mie dichiarazioni. Quindi, il medico, insieme al fiduciario, valuterà nell'attualità, se ci sono state delle innovazioni e dei miglioramenti per quanto riguarda l'attività terapeutica assistenziale, che non è detto debba essere per forza messa in essere perché potrebbe accadere anche l'inverso, colleghi senatori e senatrici.

che deve realizzarsi ed attualizzarsi l'assistenza. Se evitiamo la consultazione del fiduciario in relazione della DAT stessa, ne viene di conseguenza che si vanifica tutto.

proprio in relazione al fatto che quando si redige una disposizione di trattamento, non c'è temporalità rispetto a quella che può essere una successiva patologia e situazione clinica.

I sieropositivi hanno oggi un qualità e un'aspettativa di vita esattamente identica a chi siero positivo non è, grazie alle terapie antiretrovirali.

ha redatte possa trovarsi in uno stato anche solo temporaneo di incapacità di intendere e volere? Se fosse infatti in grado di intendere e di volere, non ci sarebbe bisogno delle disposizioni anticipate in quanto non darebbe eventualmente il suo consenso ai trattamenti che vengono proposti.

possa affermare che c'è una dichiarazione anticipata di trattamento. Poi deve esserci un fiduciario. Speriamo che l'abbia nominato e che egli si ricordi di essere un fiduciario. Quindi, ad un certo punto, il medico del pronto soccorso deve chiamare immediatamente questo soggetto che, forse

contenziosi all'infinito. Un fiduciario a un certo punto potrà dire: "Perché devo prendermi questa responsabilità? La prenda lei, signor medico, che è il medico curante di questo paziente!".

Signor Presidente, anche il mio Gruppo sottoscrive l'emendamento del senatore Romano. Faccio notare che, in realtà, quanto è stato fin qui detto evidenzia una

Perché questo stesso rigore non viene adoperato nel momento in cui la dichiarazione viene fatta? Perché questa cautela, questa precauzione svanisce d'incanto e non si prende in considerazione né un limite di tempo, di tempo, né altre garanzie, che in qualche modo possano confermare e dare valore

chiediamo che vengano inserite le parole: «e in conformità al codice di deontologia medica». Riteniamo che sia fondamentale la funzione del medico, quello che ha studiato, quello su cui ha giurato, che è il motivo per cui sta facendo quella professione: il medico come strumento di vita e non strumento di morte.

rendere ancora più forte il rapporto fiduciario tra il medico e il paziente, cosa che con questo provvedimento stiamo facendo venire meno. Di conseguenza, d'ora in avanti il rapporto tra medico e paziente sarà dato solo dalle disposizioni anticipate di trattamento su qualsiasi cosa.

e contro le *fake news* dei *no vax* o dei *free vax*, dove l'informazione veniva dettata solamente da una informazione di basso profilo scientifico a livello mediatico senza potere mai consultare il parere di un medico autorevole e competente. Stiamo facendo entrare dalla finestra, nelle DAT, con l'assenza del medico, quello che abbiamo contrastato per quanto riguarda il metodo Stamina e il tema delle vaccinazioni. Mi si dia una risposta, delle due l'una: o abbiamo sbagliato prima o stiamo sbagliando adesso.

ovviamente l'argomento non è la 5ª Commissione in sé, ma la sua notevole flessibilità, perché, poi, al comma 6, quando, al secondo periodo, si sopprime l'esenzione delle DAT dall'obbligo di registrazione e, conseguentemente, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, analoga preoccupazione non vi è stata. Quello che rileva, al di là della notevole flessibilità della 5ª Commissione, 5ª Commissione, è ciò che il senatore Romano ha sottolineato con forza, ossia il fatto che siamo in presenza di un atto che si vuole banale, banale, al punto anche da non avere un'adeguata registrazione, controfirma o pagamento delle imposte che, in questo caso, sono dovute. Più volte abbiamo contestato l'assenza del registro nazionale. Ma, al di là del rimedio che nella legge di bilancio qualcuno cercherà di porre all'esigenza di un registro nazionale, colpisce l'idea di un atto banale.

che una dichiarazione o un'affermazione, che uno fa in vita quand'è giovane e forte e non si aspetta di avere malattie in vecchiaia, possa prevalere su tutto e rendere difficilissimo uscire da una certa situazione, anche quando il medico è in grado di dire che il paziente può essere salvato. Non capisco perché vengano bocciati tutti questi emendamenti e perché qualcuno, proprio a sproposito, abbia tirato in ballo la scienza. Tutta la scienza che ha parlato qua e chi

da medico ripenso alle situazioni di urgenza. Desidererei un attimo di attenzione da parte dei colleghi della parte sinistra dell'Emiciclo, con i quali mi congratulo perché hanno trovato temporaneamente un accordo su una legge che farà molto male al Paese, ma forse bene a loro perché

del medico che non potrà pensare a cosa fare perché, nel momento dell'urgenza, non sarà libero di prendere le decisioni per il bene della persona in scienza e coscienza. Pensateci bene. Ricordo che potrebbe essere qualcuno dei nostri figli.

Signor Presidente, la logica vorrebbe che il momento di una dichiarazione anticipata, poiché dovrebbe essere un atto pensato e meditato, potrebbe avere anche una maggiore formalizzazione rispetto al momento nel quale la stessa dichiarazione viene eventualmente revocata, proprio per le condizioni di urgenza che potrebbero sopravvenire e che rendono quell'atto molto urgente e molto veloce. Il riferimento al pronto soccorso dice tutto. questa sarebbe la logica ordinaria e del buon senso. Il provvedimento in esame ha la logica inversa, e cioè quell'atto che può essere meditato e quindi anche maggiormente formalizzato viene reso scevro da qualsiasi formalità, e invece la revoca ha bisogno di due testimoni e un notaio. L'emendamento in esame non vuole capovolgere la logica, ma tende quanto meno a ricreare una simmetria

questi emendamenti hanno lo scopo di determinare una data di scadenza delle dichiarazioni anticipate di trattamento e delle loro relative disposizioni, limitandone la validità a due anni, affinché periodicamente possa esservi una riflessione su un atto così rilevante, nonostante qui si stia facendo di tutto per renderlo banale. È arrivato a fine vita anche il suo microfono, senatore lo stesso motivo per cui ha già parlato il presidente Sacconi. L'idea è di dare un tempo limite per la sottoscrizione delle DAT, in modo da permettere eventuali ripensamenti da parte del soggetto che ha sottoscritto le DAT stesse. Di conseguenza, è giusto che il tempo sia di due anni e non troppo lungo.

torniamo al tema della certezza delle dichiarazioni e all'assenza di un registro nazionale.

esistono anche momenti di conflitto fra le due Camere, che richiederebbero l'incontro dei Presidenti per dirimerlo. E questo è un caso di conflitto: sulla stessa materia, nello stesso tempo, nelle stesse ore - probabilmente o quasi - la Camera sta intervenendo perché si riconosce siffatta carenza. Vogliamo cioè che vi siano adeguate garanzie di attendibilità e di ufficialità nell'espressione delle volontà; che vi sia un'adeguata tutela della *privacy* e che

*vulnus* è veramente non casuale, come ho già detto. Siamo nella logica della banalizzazione di questo e di altri importanti atti che riguardano la vita della persona.

il quale abbiamo discusso a lungo sull'utilità di un registro nazionale, e tutti i colleghi e le colleghe dicendo che non è che non esistano altri registri; ci sono e sono previsti i registri regionali. poiché i sistemi sono interoperabili - come è noto - grazie a scelte che sono state fatte nell'ambito delle diverse leggi

Non possiamo, però, certamente dire che le DAT sono appese al nulla, perché per legge sono presso i registri regionali e, visto che

una esemplificazione chiara per tutti. Arriva un paziente che non è in grado d'intendere e di volere; il medico al pronto soccorso deve rianimarlo, perché la deontologia medica è la rianimazione, ossia fare tutto per salvare la vita alla persona.

assistito è di non essere attaccato alle macchine, di non essere riabilitato e quant'altro. A quel punto mi domando che cosa facciamo. Verrà fuori il fatto che il medico si difenderà e, quindi, aumenterà sicuramente la pratica della medicina difensiva. *(Applausi

riferiti dalla presidente De Biasi non solo non sono interoperabili - e sfido a dirmene uno che è interoperabile - ma non esistono neanche in tutte le Regioni, come non esistono altri registri, come i registri tumori. Addirittura all'interno

le basi per essere, dal punto di vista pratico, applicato nel modo giusto che il legislatore intende. Il Paese è fatto di gente reale e situazioni reali e non di quello che ci diciamo, scartoffiando di qui e di là, tra Camera e Senato, Commissione su Commissione, in fretta, svolgendo audizioni frettolose e non approfondendo

la politica è allo sbando e il senso di quello che uno deve fare qua dentro non c'è. L'ultimo giorno in cui saremo qui in Senato, e cioè l'ultimo giorno di seduta, porterò lo smalto per le unghie. Mi darò lo smalto e finalmente avrò la sensazione di aver fatto durante la seduta una cosa compiuta.

Signor Presidente, abbiamo accertato che un registro nazionale delle DAT non c'è, in attesa che si possa dar luogo all'approvazione dell'emendamento alla Camera. Quindi, mi devo attenere al testo che stiamo valutando e approvando o meno.

significa che non tutte le Regioni sono obbligate: alcune le adottano, altre no. Se non è un obbligo l'adozione, ne deriva come conseguenza che la rete nazionale non può esistere. Faccio un'ulteriore riflessione finale e questa - devo dire - è una chicca del comma 7, laddove si dice che bisogna depositarle nell'ambito di un fascicolo, di una banca dati, laddove c'è - e laddove non c'è? e poi si dice anche «lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili».

di poterle non solo pubblicare, ma anche di renderle immediatamente accessibili a chi vuole intervenire sempre e soltanto nell'interesse del paziente.

Grazie

credo di riprendere un discorso ben noto che ho già illustrato in sede di discussione generale. Esiste una sostanziale differenza tra disposizione e dichiarazione: la relazione di cura si realizza solo con la dichiarazione, mentre la disposizione è contraddittoria a qualsiasi forma di relazione di cura. La disposizione è imperativa;

ci sono anche il codice deontologico e i vari pareri del Comitato nazionale per la bioetica. Se relazione di cura c'è, c'è solo la dichiarazione; se non c'è relazione di cura, allora dobbiamo cancellare il comma 2 dell'articolo 1 e modificare anche l'articolo 5, che parla di pianificazione condivisa delle cure. Ancora una volta devo dire che c'è una contraddittorietà tra quello che è il principio di riferimento e il richiamo legislativo che non concretizza assolutamente.

verrà bocciato, ma mi rimane una sorta di soddisfazione per aver testimoniato da questa mattina quello che è l'interesse prioritario del paziente, senza accanimenti e senza abbandoni, nella proporzionalità delle cure. Grazie per l'attenzione che mi avete riservato.

che parla di differenza sostanziale tra dichiarazione e disposizione. Ormai lo abbiamo detto in tutte le salse e non so più neanche in quale lingua dirlo:

per ricordare che la nostra proposta emendativa vuole esplicitare che è fatta salva ogni valutazione del medico in ordine a circostanze non considerate o sopravvenute rispetto alla pianificazione delle cure condivise.

in dichiarazione di voto per motivare il no all'articolo 5. Anche su questo articolo, intitolato alla pianificazione condivisa delle cure, è stato sistematicamente e cinicamente, per ordine editoriale ricevuto da quelli che devono scrivere «fatto», deciso di respingere qualsiasi emendamento. Questo ci lascia, francamente, esterrefatti. Penso agli emendamenti che ipotizzavano la possibilità di cure sopraggiunte, in quanto la medicina ha una evoluzione, e quindi la possibilità di aggiornare le decisioni e di rivederle rispetto a dichiarazioni, peraltro con meccanismi macchinosi che vedo qui evocati, come le videoregistrazioni. Quanti, poi in concreto lo faranno? Quanti margini di incertezza lascerà questa legge?

C'è un problema di ricandidature? C'è il problema che il gruppo editoriale «X» non ti mette la foto e non ti candida, visto che c'è una difficoltà di spazi? Un tema di questa natura non andava trattato in queste circostanze, con queste modalità e con questo cinismo. È una vergogna che ricada sul Senato averlo trattato in questa maniera, con tutte le contraddizioni che anche questo articolo comporta, per non aver voluto migliorare le normative riguardanti il comportamento dei medici,

alla fine di questo articolo, non vediamo venire meno le ragioni per le quali abbiamo sostenuto moltissimi emendamenti.

coraggiosa e coerente, con la quale ha fatto di tutto per proporre alleggerimenti alla rigidità di questo disegno di legge. La rigidità di questa legge sta nell'essere stata proposta *ne varietur*. Questa mattina, con una certa eleganza, mi pare un altro senatore del centrosinistra, il senatore Bianco, ammoniva alcuni di noi a non introdurre la cura di Stato. Facciamo nostra questa preoccupazione, però ci sarebbe piaciuto che almeno su un emendamento ci fosse stata, da parte dei colleghi del centrosinistra, la preoccupazione di un eccesso di eticità della rigidità della vostra proposta normativa. Capiamo tutte le ragioni volte a portare a casa il risultato, alle nostre ragioni di opposizione. Voi dite che confinano con l'ostruzionismo. Certo, nell'opposizione di merito a un provvedimento si arriva alle soglie dell'ostruzionismo, ma il comportamento che fin dalla discussione generale è stato tenuto in quest'Aula da parte di quei colleghi che non hanno ritenuto il lavoro del Parlamento, in questa circostanza, degno di un loro contributo

Grazie,

Entra in vigore una normativa e c'è questa transizione di dichiarazioni fatte in un'altra epoca e in un altro contesto, forse senza avere nemmeno la consapevolezza di quanto diventino vincolanti quelle dichiarazioni. Uno ha fatto una dichiarazione dieci anni fa presso un notaio non pensando di mettersi in un meccanismo infernale come questo, con i figli che votano e i cugini e nipoti intorno al

averlo letto - dice che ciò che è stato scritto prima in un altro contesto viene trattato con le procedure di questa nuova legge, che sono quelle che abbiamo illustrato. Ecco perché si chiede con emendamenti dei vari Gruppi la soppressione di questa norma

all'approvazione di un testo senza che questa Camera l'abbia potuto esaminare nel dettaglio attraverso un confronto tra le diverse culture politiche, in assenza totale di un confronto, ma ci consenta almeno di sottolineare, e credo che anche il compagno Quagliariello abbia il diritto e dovere di farlo.

Lei sa che non sono mai intervenuto se non in ragione di un emendamento presentato, come in questo caso. Parlo anche per gli emendamenti successivi, che sono sostitutivi del comma 6; faccio, quindi, questa dichiarazione anche per i futuri emendamenti. Come ha detto poco fa il collega Gasparri, siamo in presenza di una norma transitoria che non ha precedenti e che conferma la volontà di banalizzare questa dichiarazione. Addirittura si danno gli stessi effetti di cui al presente provvedimento ad atti depositati presso un municipio in passato.

di tutti quei caratteri di pubblicità e di riservatezza che una dichiarazione così rilevante dovrebbe avere. Molto meno che vendere un motorino usato. innanzitutto, per fatto personale vorrei chiederle un giurì d'onore, perché sono stato definito «compagno»; io ho anche qualche problema con la definizione di «cittadino», che richiama la Rivoluzione francese,

Anche in questo l'anagrafe non aiuta. Signor Presidente, devo dirle sinceramente che sull'articolo 6 prenderemo la parola più di una volta in tempi congrui, ma questa è una battaglia di testimonianza e non credo che abbiamo approfittato della sua cortesia e di quella dell'Assemblea. Penso che questo sia un comportamento di serietà per chi ha delle opinioni che contrastano con questa legge e che vuole evidenziare la sua fondamentale non serietà.

delle dichiarazioni antecedenti che sono state lasciate presso il Comune e presso i notai non è serio. Ciò soprattutto per due ragioni: queste dichiarazioni possono non rispondere a quanto è previsto in questa legge; in secondo luogo, perché rendono ancora più difficile quel pasticciaccio brutto dei registri differenti. ma sarebbe il caso di chiamare qui il Ministro della salute e chiedere se veramente ritiene che sia possibile fare un registro nazionale che segua quanto previsto e con la cifra stanziata nell'attuale legge di stabilità. Questa norma si presta ad ulteriori equivoci.

i provvedimenti precedenti. Signor Presidente, sono queste le ragioni per le quali chiediamo la soppressione dell'intero articolo.

quindi oggi pomeriggio, la notturna e la prima parte della seduta di domani, fosse riservata a chi volesse intervenire. Questo è stato detto nella Capigruppo e quindi credo che noi stiamo esercitando il nostro diritto di motivare degli emendamenti su una questione estremamente seria.

iniziative totalmente estranee e fuori dalla legge, di tipo propagandistico, per invitare i cittadini a consegnare presso i Comuni queste dichiarazioni di fine vita. Come sono state depositate? Con che spirito sono state depositate? Erano una testimonianza? Cosa c'è scritto dentro a quelle disposizioni? Erano fatte nell'ottica di preoccuparsi in un futuro di essere soggetto o oggetto di cure mediche, o eravamo all'interno una campagna pubblicitaria e propagandistica per spingere il Parlamento ad assumere determinate posizioni? Con questa sanatoria si dà a tali iniziative propagandistiche la dignità che dovrebbe avere invece un documento dal quale dipende la vita futura di una persona. Capisco bene che anche i nostri emendamenti, che volevano in qualche modo non solennizzare ma rendere credibile anche il momento in cui queste disposizioni venivano dettate, sono stati bocciati; un conto è fare una disposizione a legge vigente, con tutti i punti interrogativi che ci sono e rimangono su dove vengono depositate (nel registro nazionale o in quello regionale) e un conto è stabilire che in 8.000 Comuni italiani possono essere state depositate

l'imperativo categorico era che non si modificava niente perché il provvedimento non doveva tornare alla Camera, anche le incongruità più incredibili rimangono, ma rimangono come una vergogna per chi le approva. infatti vedere domani, quando usciranno quei trattati critici sulla legge fatte dai vari istituti giuridici che andranno ad approfondire questi punti, cosa scriveranno di norme di questo tipo: a quale tipo di codice civile, di procedura civile, di diritto costituzionale, di pandette romane si rifaranno per far entrare in vigore disposizioni private depositate un bel giorno presso qualche Comune.

perché domani mattina, visto l'andamento dei lavori, le dichiarazioni di voto si svolgano alle ore 9,30 senza attendere le ore 11. Pertanto, se non comunicate con i vostri Capigruppo, io non sono in grado di mantenere o rispettare i tempi. Senatore Gasparri,

Questo emendamento dice che i documenti fatti nel passato sono nulli all'entrata in vigore di questa legge, che è esattamente il contrario di quello che dice la norma transitoria. ripeto le motivazioni, come ho diritto di fare, pacatamente e ragionatamente, senza che qualcuno me lo debba impedire: è sbagliato giuridicamente traslare nell'epoca nuova, con effetti diversi, con cogenze diverse, con obblighi diversi, con automatismi diversi, cari colleghi, una dichiarazione fatta in un altro contesto. È vero che in quest'Assemblea abbiamo anche sancito la retroattività delle norme penali. Questo si può dire o devo chiedere un permesso speciale? Abbiamo assistito vicende storiche, in cui il voto segreto si è concesso o non si è concesso a seconda delle convenienze o in cui alcune leggi penali sono state applicate retroattivamente. Qui siamo all'applicazione futuribile della dichiarazione retroattiva che una persona ha fatto in un altro contesto, in cui la poteva cambiare, stracciare non aveva alcun valore giuridico perché, non essendoci la legge, la persona che ha fatto una dichiarazione in passato, l'ha fatta per una sua autonoma volontà, senza alcuna consapevolezza della rigidità e dell'obbligo che la legge nuova, che allora non c'era, avrebbe determinato. È un po' lo stesso ragionamento della retroattività della norma penale, che non si può sancire; qui siamo alla futuribilità della norma sulla dichiarazione, che viene messa e inscatolata in un contesto diverso. È molto grave questo fatto, Presidente, dal punto di vista morale, etico e giuridico ed è una questione che vi dovreste porre e quindi dire che sono nulle le cose dette prima. C'è un regime diverso e uno fa una dichiarazione sapendo che si mette dentro questo circuito infernale del medico che non conta e dei parenti che votano intorno a letto. Lo so che dà fastidio ad alcuni che si dicano queste cose, ma sono le pure e semplici verità. Questo emendamento azzererebbe il contatore: il regime giuridico è diverso e chi fa la dichiarazione, se la vuol fare, sa che si infila in questo *tunnel*, in cui non deciderà più niente lui o nessun

una dichiarazione fatta senza sapere che c'erano tutti questi vincoli. È una follia! Io mi auguro che siano pochissime le dichiarazioni, perché poi il bello di queste leggi è che vengono invocate da molti, ma poi vengono usate poco (basta andare a vedere quelle sulle unioni civili o altre leggi quanto siano state Quindi, voi fate delle leggi per pochi che sono anche sbagliate. Credo che se una legge è giusta, vada fatta anche per uno; se è sbagliata ed è per pochi, credo che questa sia una motivazione per votare ancora più convintamente a favore di questo emendamento.

Signor Presidente, credo che su questo argomento si debba insistere, sperando che qualche esponente della maggioranza - non dico il Governo, che si è rimesso all'Assemblea - o qualcuno che dice che la scienza va rispettata, anche quella giuridica, si alzi e abbia la buona fede di dire: vogliamo assolutamente approvare questa legge e quindi anche le disposizioni completamente fuori senso e fuori logica giuridica le approviamo così come sono,

la dichiarazione di voto sull'articolo 6 è ovviamente coerente con quanto abbiamo avuto modo di dire in fase di illustrazione degli emendamenti, purtroppo non approvati. Voglio che resti agli atti che, con questo articolo 6, si dà una vigenza futura a volontà rese in un momento in cui - per chi le avesse realmente rese e la norma si riferisce a questa ipotesi

certo modo, ma non c'è stata poi mai una prova, scritta o video. Questa è la storia italiana, che abbiamo anche discusso in quest'Aula. Ve lo ricordate o no? Siamo andati all'interpretazione retroattiva di un'affermazione forse fatta in un paradosso, come dire: stasera ho mangiato troppo e mi sento di morire, non mi soccorrete perché voglio esplodere. persona può dire qualsiasi fesseria in ogni momento. Qui invece siamo di fronte alla trasposizione in un regime nuovo di dichiarazioni fatte in assenza di vincoli e legami: è un obbrobrio giuridico e morale e questo resta, anche se lo approvate. Queste cose saranno poi tritate - spero - in altre sedi giuridiche dal giudice delle leggi, da chi deve verificare. Pertanto, voto convintamente contro l'articolo 6,

sulle bizzarrie giuridiche del Senato, su cui gli specialisti della materia si potranno non dico divertire, ma impegnare molto. Ribadisco quindi

Quel che non ci convince dell'articolo 6 è il frutto della lunga discussione che iniziammo la scorsa settimana. In particolare, però, voglio effettuare

del documento che dispone in merito al trattamento sanitario l'abbiamo già fatte e hanno una forma di eternità e immodificabilità che che nessun'altro documento nell'ordinamento giuridico italiano si è mai visto attribuire. E c'è la preoccupazione di ribadire come si possa andare anche da un notaio. State attenti, colleghi della sinistra, voi che siete tanto sensibili al liberismo del professor Giavazzi, arriverà il consueto articolo contro i notai, valorizzati da questo

Inoltre, non sono mai stato un entusiasta del federalismo quanto l'ottimo Presidente della nostra seduta, ma questo federalismo dispianantesi su più di 8.000 Comuni in materia di vita e morte mi fa pensare che, benché stonato nei tempi, nei modi e nelle procedure, quel tentativo di aggiustare la frittata attraverso l'istituto regionale, da me ancor meno amato di quello comunale, abbia un suo fondamento. Dispiace, però, che questa sovrapposizione di tempi, modi e procedure fra Camera e Senato

PLI))*. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 prevede la soppressione dell'articolo 7, che stabilisce la clausola di invarianza finanziaria. Ora, né nella versione disomogenea e confusa dei registri regionali, come previsto nel testo in discussione, né nel caso in cui si istituisca un registro nazionale, così come previsto dalla legge di bilancio in discussione nell'altro ramo del Parlamento, è possibile che l'applicazione di queste norme non comporti maggiori oneri per le casse dello Stato. Questo è talmente vero, signor Presidente, da essere confermato proprio attraverso l'inserimento e l'approvazione di un emendamento nella legge di bilancio che istituisce un fondo di 5 milioni di euro per la gestione del del registro nazionale. Questi 5 milioni non saranno sufficienti, ma stabilire che una legge di questa complessità, con questi problemi, possa essere applicata in invarianza

che penso possa essere utilizzata anche per rivalutare parte del lavoro che abbiamo compiuto e che ha visto come motivazione di riferimento in molte delle citazioni fatte dai colleghi che si sono opposti a questa norma il fatto che si tratti di una norma fatta male. Perché è una norma fatta male? Intanto perché molto di quello che viene presentato come una novità è invece un già visto: già oggi esiste la disciplina adeguata sul consenso informato, come confermato dalla

quest'Assemblea, riguardano, per esempio, l'eliminazione dell'obiezione di coscienza del medico, la sostituzione della professionalità medica con un ruolo tracimante, ancora una volta, della magistratura, un'incidenza fuori dalla misura nei confronti del ruolo dei familiari e - come già stato più volte ripetuto un attacco sistematico a quella che possiamo definire l'alleanza terapeutica. Insomma, una concezione di marca illiberale. Le riflessioni proposte quindi, di coloro che considerano la norma un passo avanti di civiltà, sono in realtà da ribaltare proprio alla luce di questa semplice considerazione: c'è dietro una concezione dello Stato per cui lo Stato è tutto e la persona è niente. In questo senso, gli emendamenti di natura soppressiva hanno la funzione di arginare siffatto modo di ragionare.

l'assurdità dell'invarianza degli oneri di finanza pubblica, che qui viene disposta. Il collega Quagliariello ha ricordato poco fa il fondo che, contemporaneamente, è stato inserito nella legge di bilancio alla Camera dei deputati, a dimostrazione del fariseismo con cui è stato scritto l'articolo Grazie, voluti dalla maggioranza e, ancor più, quando si tratta di provvedimenti divisivi a forte contenuto ideologico. Allora, tutti gli argini di finanza pubblica vengono meno e la disponibilità a a letture molto duttili dell'eventualità degli oneri di finanza pubblica consente di superare ogni problema di copertura. La sottolineatura che faccio va soltanto a confermare la protervia di una linea ideologica, che non ha mai cercato soluzioni nel segno della composizione delle delle diverse culture politiche e la determinazione con cui è stato perseguito l'obiettivo di una legge fortemente divisiva, perché tale sarà, soprattutto nella società.

quasi si fosse profeticamente previsto quello che sarebbe successo alla Camera dei deputati, proponevano di escludere dal blocco delle spese, cioè dall'invarianza di spesa che l'articolo 7 proclama

come vedete, potremmo farle anche stasera le dichiarazioni di voto finali. Perché non farle? Alle 21,30 sarebbe tutto finito, così «la Repubblica» domani potrebbe uscire con la "targhetta" giusta.

possano uscire con la notizia. Quindi, non c'è alcuna attività dilatoria. C'è piuttosto una attività di illustrazione delle motivazioni che valgono anche per l'articolo 8, perché sono stati respinti gli emendamenti

nel futuro ci saranno probabilmente contese, perché i figli messi in minoranza, intorno al letto di morte, dalle votazioni familiari che avete previsto con questo provvedimento, potranno fare ricorsi, istanze, non so a chi. Qualcuno si troverà: un ricorso non si nega a nessuno.

legge nel suo complesso sono molteplici: gli errori, gli strafalcioni giuridici, le aberrazioni di ordine etico e morale, viste sotto un profilo di assoluta laicità; ancora, le violazioni ai principi di deontologia dei medici, le pressioni sulle decisioni che le strutture sanitarie dovranno prendere, l'impedimento dell'obiezione, il conformismo dilagante. Ci sono realtà minoritarie che riescono a imporre leggi sbagliate invece di lasciare spazio all'alleanza terapeutica, alla saggezza delle famiglie, alla competenza dei medici, a quello che deve essere il decorso naturale delle cose, perché, poi, l'obiettivo sarà quello di arrivare all'eutanasia. Nel prossimo Parlamento non ci sarà, credo, una maggioranza per l'eutanasia, quindi chi pensava, con questo disegno di legge, di fare il primo tratto di strada verso una definitiva deriva e affermazione eutanasica, troverà l'impedimento delle elezioni, che, capisco, qualcuno vorrebbe protrarre al 2054, ma i cinque anni sono pressoché scaduti. Non so se, come ha scritto «la Repubblica» si si voterà il 4 marzo, ma tanto qui siete una redazione distaccata di quel giornale, quindi anche la data sarà buona. Il prossimo Parlamento certamente non potrà portare a ulteriori conseguenze questo modo errato e assurdo di legiferare, del quale chi ha voluto farsene vanto si assume la responsabilità, ma proprio sotto il profilo della giurisdizione, non sotto altri profili, che ciascuno discuterà in altri ambiti con la propria coscienza. Per questo, annuncio il voto contrario sull'articolo 8, giudizio

e non scoprire le cose solo in Aula, certe perle che emergono anche alla fine dell'articolo 8 sarebbero emerse precedentemente. Per l'esperienza che ho io (e un po' ne ho) dei rapporti con il Quirinale, con le procedure parlamentari e con i tempi che servono affinché una legge sia pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, ben difficilmente questa legge andrà in *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore

dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, per avere una qualche informazione sulla sua applicazione: quattordici mesi, perché andiamo all'aprile del 2019. Lo stesso vale Le Regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno e, poiché questa legge entrerà in vigore all'inizio del prossimo anno, delle Regioni ne parleremo un anno dopo. Quindi, approviamo una norma, che magari applichiamo anche al Ministero della giustizia (e per tali per i quali l'applicazione della legge nei mesi più importanti sarà sconosciuta al Parlamento. Gli adempimenti del Ministero della salute e gli adempimenti delle Regioni, infatti, vengono proiettati in un tempo incredibilmente lontano. Si poteva rimediare. Era una delle tante cose che potevano essere aggiustate in Commissione, dove l'ostruzionismo lo ha fatto la maggioranza. Se la maggioranza, infatti, avesse detto che era disponibile ad accettare, ad esempio, il termine «dichiarazione» invece che il termine «disposizione» e altre due o tre modifiche delle parti più aberranti e incomprensibili di questa legge, si poteva benissimo concludere un accordo. Ma poiché, fin dal primo minuto, è stato chiaro che la maggioranza non voleva cambiare assolutamente nulla di questo testo, totalmente sbagliato e per certi aspetti grottesco, il risultato è - e per questo l'Aula serve e lo vedremo dopo, quando parleremo della della modifica del titolo - che è emersa tutta una serie di incongruenze, una dietro l'altra, che hanno mostrato la debolezza assoluta di questo testo. mi associo alle considerazioni svolte, soprattutto dal collega Gasparri, a proposito della utilità di una relazione anche del Ministero della Giustizia. Lasciamo, quindi, questa considerazione alla alla valutazione della prossima legislatura, quando mi auguro si vorranno monitorare con attenzione gli esiti di questo provvedimento, non solo dal punto di vista sociosanitario (e certamente questo profilo è rilevante), ma anche dal punto di vista giurisprudenziale. Con ogni probabilità, infatti, si determinerà contenzioso, si produrranno abusi che potrebbero integrare fattispecie penalmente rilevanti, si potrebbero determinare anche azioni di responsabilità civile nei confronti dei medici. Temo che il provvedimento produca questi esiti anche in ragione della sua ricorrente debolezza tecnica, frutto proprio di un approccio rigido, ideologico, chiuso ad ogni confronto, che ha fatto sì che si sia svolta questa triste pagina parlamentare, fatta di monologhi che solo raramente hanno avuto interlocuzione, nonostante le modalità di esame del disegno di legge non consentissero certo l'esercizio di una attività ostruzionistica. Ciononostante, ripeto, il confronto non si è svolto. Ho visto molti colleghi accingersi a votarlo e condividerlo, però mi è parso con un certo imbarazzo, soprattutto alla luce di quelle convinzioni che so essere anche loro e che, in questo caso, sono state sottomesse a una "ragion politica" e o meglio "ragion partitica",